finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Casini. A questo punto, visto che abbiamo un attimo di riflessione temporale, ritiriamo tutte le tessere cui non corrisponde la

Colleghi, non intendo aprire un dibattito su pasticcini, caffè e altre cose. Il Presidente ha dato lettura della sua interpretazione e delle precedenti interpretazioni della Giunta per il Regolamento. La sede competente non è la Conferenza dei Capigruppo, ma sarà la Giunta per il Regolamento, ovvero il Consiglio di Presidenza, a decidere eventualmente in maniera differente. Fintanto che c'è quel pronunciamento del Presidente intendo applicarlo

(testo 2) per dire che finalmente, dopo una discussione che è durata molto tempo, abbiamo condiviso l'opportunità di utilizzare questa circostanza per poter rimediare ad un *vulnus* che si era determinato all'interno del Copasir, perché, in virtù dei movimenti politici di questi mesi, il partito di Forza Italia non aveva più un rappresentante all'interno organismo. Questo ovviamente, essendo Forza Italia, non soltanto una forza politica molto rappresentata in Parlamento, ma anche un partito che si è candidato alle elezioni e ha eletto i propri rappresentanti parlamentari, mi sembrava assolutamente Abbiamo immaginato di farlo attraverso questo emendamento, che mi auguro peraltro possa essere condiviso unanimemente da tutta l'Assemblea, anche perché questa è una discussione che abbiamo più volte svolto

pur condividendo in linea di principio il fatto che al Copasir siano rappresentate tutte le forze politiche, il Comitato ha in realtà una una conformazione che è data da cinque senatori della maggioranza e cinque dell'opposizione. Non sono rappresentati i partiti singolarmente, ma viene rappresentata la maggioranza e l'opposizione. Viene fatta un'istantanea ad inizio legislatura (in ottemperanza a quanto prevede la legge n.

In linea di principio accetto che la minoranza venga potenziata in seno al Copasir (e quindi ci asterremo su questo emendamento), ma non trovo corretto che venga scelta questa via di legiferare a tempo determinato, fino alla fine della legislatura,

per alterare la composizione di un Comitato così importante e così delicato.

Presidente, il voto dei Conservatori e Riformisti, come già avvenuto in Commissione, è certamente favorevole al provvedimento, perché finalmente si mette chiarezza e che si è dovuto votare, spesso con urgenza, senza regole fisse e certezze per i nostri militari impegnati all'estero. Finalmente si pone un quadro normativo chiaro, che definisce ruoli e competenze a tutti i livelli e, innanzitutto, garantisce i nostri militari nell'azione che svolgono, per il bene delle comunità in

che spesso non sono affatto chiare e mettono i nostri militari nelle condizioni meno adatte per affrontare i pericoli, come spesso è accaduto anche a forze dell'ONU. Spesso si assiste infatti a massacri, ma le regole di ingaggio prevedono che non si possa intervenire. Le regole di ingaggio devono essere chiare,

cercare di non diventare subalterni a nessun'altra forza politica mondiale; «subalterni» non è un termine usato a sproposito, anche perché dalle primavere arabe in poi c'è stato un appiattimento della politica estera e militare nazionale sulla politica estera e militare americana. Ci è stato imposto di liberare il Nord Africa dai dittatori e di dare libertà a quei popoli; è stato svolto un intervento militare importante in Libia e infatti abbiamo dato la libertà a quei popoli: la libertà di morire di fame.

La nostra fortuna è che nel mirino americano doveva esserci anche la Siria ma l'intervento russo ha evitato che il disastro fosse generalizzato. Oggi gli americani ci chiedono

prima che scelte sciagurate di subalternità ancora una volta verso Paesi d'oltreoceano ci portino in un conflitto con mille risvolti tra i più imprevedibili. il testo delle disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali. Esso prevede una nuova disciplina di autorizzazione delle prossime gestioni, ma soprattutto toglie un aspetto che ultimamente era intollerabile, cioè il totale arbitrio del Governo nelle politiche di stabilità internazionale. I vari

Si stabilisce che potremo partecipare a missioni sovranazionali, qualora istituite sotto l'egida di organismi riconosciuti come l'ONU, la NATO, l'OSCE e l'Unione europea.

sottosegretario Alfano, non porterà lei pena di quello che sto dicendo, ma il Governo deve darne notizia alle Camera alle Camera e non nei *talk show*. Noi abbiamo visto il presidente Renzi annunciare ciò che intende fare in materia di intervento militare, non alle Camere (luogo deputato a stabilire se autorizzare o no), ma addirittura ridendo e scherzando, tra giochi, in

Una cosa buona è ciò che si farà con l'istituzione della sessione parlamentare completamente dedicata all'andamento delle missioni. Vorrei ricordare quel tanto o quel poco che ha fatto la Lega, che ha contribuito su questo argomento laddove, proprio a tutela dei nostri soldati, ha chiesto di inserire nel capo IV, che regola le disposizioni penali, che i nostri soldati siano soggetti non al codice penale militare di pace, ma al codice militare

di diverso rispetto a conflitti veri e propri. Siamo soddisfatti del fatto che si ripristini un po' l'ordine costituzionale, anche perché, dopo tutte le riforme che sono state portate in quest'Aula, abbiamo visto un eccesso di concentrazione di poteri sul Governo e sul Presidente del Consiglio, che non sono consoni ai dettami di una Costituzione che possa definirsi ancora democratica. Un solo partito vincerà le elezioni; un solo partito governerà il Paese; un monocolore di Governo sarà destinato a governare l'Italia; quella maggioranza che si forma nel *post*‑elezioni sceglierà tutte le alte cariche della magistratura; avrà la possibilità di appianare ogni processo evolutivo; avrà la possibilità di nominare un proprio Presidente della Repubblica e nominerà tutti i vertici del sistema radiotelevisivo (direttori di rete e di testata). Controllo della magistratura, controllo delle alte cariche dello Stato, controllo del sistema dell'informazione; ci mancava anche che il Presidente del Consiglio potesse

tramutando sempre più in quello che era il sistema romano, che da consolare diventava dittatura, ma allora era giustificato dai momenti di difficoltà;

dell'acquisizione nel nostro Paese di una vera e propria cultura della difesa. Il fatto di non delegare continuamente a meccanismi provvisori l'autorizzazione delle missioni di pace all'estero è oggettivamente un passo in avanti per quella che noi chiamiamo la cultura di difesa. Mi auguro, peraltro, che a questa norma possano collegarsi quei provvedimenti che consentono di tornare a riflettere in modo adeguato sul tema degli investimenti e dei costi d'esercizio del sistema della difesa. Inevitabilmente, infatti, non si sarà mai pronti al momento giusto se per tempo non si sarà potuto pianificare pianificare l'impianto di difesa del nostro Paese e la rete di difesa che deve essere predisposta nel nesso con gli alleati sia sul piano europeo che sul piano occidentale.

cioè la norma che ascrive alla Presidenza del Consiglio la possibilità di conglobare le risorse di *intelligence* e quelle di alcuni reparti speciali della Difesa per i provvedimenti di urgenza, laddove lo si reputi necessario, a difesa degli interessi nazionali. Questo è un provvedimento che collegando le risorse di *intelligence* a quelle dei nostri corpi speciali rende sicuramente un buon servizio, non solo alla cultura della difesa ma anche alla provvida operatività del nostro Paese.

amministrazione. Delegare alla Presidenza del Consiglio ciò che non si crede essere in grado di inquadrare in termini precisi ed esatti

diventata più che un organo di coordinamento un vero e proprio tappo per la pubblica amministrazione. Con questa mia considerazione intendo fare un ultimo rilievo: che sia il luogo sbagliato è testimoniato dal fatto che proprio la Presidenza del Consiglio è la fonte attraverso la quale siamo venuti a conoscenza, grazie alla stampa, di un livello di provvedimento che doveva rimanere segretato,

perché o ci convinciamo di dover cambiare la Costituzione in modo che possa essere supportata la natura del provvedimento stesso o è bene che si torni ad una consuetudine di percorso che, pur garantendo la piena organicità nell'operato di *intelligence* e corpi speciali,

il provvedimento. Si tratta, infatti, di una legge attesa da anni visto che attualmente il quadro normativo in merito è stabilito da singoli decreti contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e del relativo finanziamento; un aspetto non da poco perché, grazie a questo disegno di legge, l'Italia uscirà da quella gestione emergenziale a causa della quale i nostri militari spesso hanno rischiato di rimanere privi di copertura dal punto di vista assicurativo ed economico, anche nel corso delle missioni. missioni. Le operazioni militari in zone di guerra caratterizzano ormai il ruolo italiano nella politica internazionale, principalmente nella lotta e nella prevenzione del terrorismo. In questo senso riveste un'importanza notevole il capo V della legge aggiunto qui in Senato, che prevede, all'articolo 19, «Disposizioni in materia di *intelligence*» per l'adozione di misure di contrasto, in situazioni di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero. A questo proposito non possono non venirci in mente gli attentati di Parigi. La lotta al terrorismo, purtroppo, non è una battaglia che possiamo scegliere o decidere di non combattere. D'altro canto, però, secondo l'articolo 11 della nostra Costituzione: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

per mantenere questa pace siamo impegnati in una trentina di missioni con circa 4.500 uomini. Il nostro Paese è il settimo contributore al bilancio ONU e la nostra partecipazione è particolarmente apprezzata soprattutto grazie all'enorme capacità di dialogo dei nostri contingenti. In questo senso, il disegno di legge prevede la partecipazione alle missioni dei corpi civili di pace, un contingente sperimentale costituito da 500 giovani volontari nell'ambito del servizio civile nazionale, e intende valorizzare il ruolo delle donne nella costruzione della pace al livello internazionale. Sul fronte economico, le polemiche sorgono spontanee quando si parla dello stanziamento dei fondi per le missioni internazionali in tempi di crisi e di difficoltà economiche. Argomenti assolutamente giusti e condivisibili se non fosse che, garantire la pace al livello internazionale e sedare i conflitti in zone del mondo dove la democrazia non è compiuta oltre ad essere un'azione eticamente giusta risponde anche al nostro specifico interesse di cercare di frenare sul nascere gli estremismi che nel corso degli anni, e purtroppo ancora oggi, hanno minacciato e minacciano gli equilibri occidentali, da Al Qaeda all'ISIS. Fenomeni drammatici che mettono a rischio le popolazioni dei Paesi del Medio Oriente, rallentando lo sviluppo dei processi di modernizzazione che molti di questi Stati stanno faticosamente cercando di portare avanti, ma anche la nostra sicurezza. missioni che l'Italia deve mantenere cercando di farlo nel migliore dei modi. E questo provvedimento traccia proprio i confini per operare con metodo seguendo il modello più giusto. Lo fa prevedendo un processo decisionale che coinvolge il Governo, il Presidente della Repubblica e il Parlamento per l'autorizzazione delle missioni: si parte da una delibera del Consiglio dei ministri che viene adottata, previa comunicazione al Presidente della Repubblica, con l'eventuale convocazione del Consiglio supremo di difesa, e poi trasmessa alle Camere. Le comunicazioni del Governo dovranno essere molto dettagliate e comprendere anche l'individuazione della disciplina penale applicabile alle singole missioni. Un processo che non terminerà comunque con l'autorizzazione della missione da parte del Parlamento, ma proseguirà con una relazione analitica annuale che il Governo dovrà presentare alle Camere ogni anno, entro il 31 dicembre. Mi sembra che questo rappresenti anche la giusta valorizzazione del ruolo del Parlamento. Infine, sul fronte economico si prevede di istituire, nello stato di previsione del MEF, un fondo *ad hoc*, sostitutivo di quello già esistente, destinato alle missioni in cui confluiscono anche le risorse per le politiche di cooperazione e gli interventi per il sostegno dei processi di pace. E ancora: vengono stabilite le indennità di missione e il trattamento assicurativo dei militari, si affrontano le ipotesi di prigionia, si prevedono orari di lavoro, riposi, e si istituisce la figura del consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale, proprio al fine di rafforzare questo ruolo di costruttori di pace e di avvicinamento con i civili che contraddistingue l'azione italiana. Si tratta, dunque, di un provvedimento puntuale e preciso che non lascia nulla al caso. Un primo passo fondamentale che sottrae un tema cosi importante alla decretazione d'urgenza, affrontando con serietà una problematica complessa. L'Italia è sempre stata in prima linea nella difesa della democrazia e della pace e continuerà ad esserlo. Da oggi, abbiamo anche quest'arma in più.

la discussione in Aula è iniziata il 15 settembre. Ieri, dopo circa sei mesi, abbiamo iniziato a votare gli emendamenti. Io penso che temi di questa portata, quando parliamo di sicurezza nazionale, che dovrebbero indurci ad esprimere un voto unanime o il più ampio consenso, proprio per dare più forza a quanto ci accingiamo a votare, debbano avere un *iter* legislativo serio. E io auspico che temi di questa dimensione e di questa rilevanza abbiano un percorso serio. Entrando nel merito del provvedimento al nostro esame, al di là di ogni strumentalizzazione politica, esso è meritevole d'attenzione, precisione e concretezza. Pensiamo che sia giunto il momento che il nostro Paese si doti di uno strumento legislativo generale stabile, preciso ed ordinato. In una situazione internazionale in continua evoluzione, una legge quadro organica che disciplini il nostro intervento nelle missioni internazionali e gli interventi di cooperazione, non solo è necessaria ma è, addirittura, indispensabile per fornire una cornice normativa unitaria, organica e strutturata. Ne consegue, quindi, una più rapida azione di deliberazione, fermo restando la responsabilità che l'Esecutivo ha di fronte al Parlamento ed al Paese. Uno degli aspetti più interessanti del provvedimento è che spetterà al Consiglio dei ministri la delibera in ordine alla partecipazione italiana ad una missione internazionale, che dovrà poi essere comunicata al Presidente della Repubblica e successivamente alle Camere, per ricevere l'eventuale autorizzazione definitiva. Questo procedimento, che da alcuni può essere visto come un eccesso di potere del Governo, in verità altro non è che l'individuazione in termini concreti di coloro che si occupano fattivamente di questioni specifiche, all'interno di un quadro geopolitico fortemente in evoluzione. Mi preme sottolineare l'importanza delle disposizioni in materia di *intelligence*, già oggetto dell'esame di quest'Aula nell'ultimo decreto di proroga delle missioni internazionali (articolo 7-*bis*), che abbiamo stralciato dal presente Siamo oggi di fronte a scenari dove la sola strategia militare non basta più. Per una serie di variabili come la globalizzazione, l'informatica, la finanza internazionale e così via, si è passati a una vera e propria rivisitazione del concetto di sicurezza e, conseguentemente, dello stesso concetto di *intelligence*. Con le mie proposte emendative avevo cercato di porre l'attenzione sul tema dell'utilizzo dei dati biometrici da parte del personale militare impegnati in sede operative. Auspico che il Governo prenda in considerazione in una prossima occasione la materia, poiché investire in *intelligence* significa anche questo, ovvero operare in maniera preventiva con la raccolta dei dati. A tal proposito, cito quanto ho avuto modo di sentire dal coordinatore dell'antiterrorismo dell'Unione europea Gilles de Kerchove, che sottolineava l'impegno delle nuove frontiere tecnologiche, che ci permettono, oltre al riconoscimento delle impronte digitali, anche il riconoscimento facciale. La considerazione delle minacce non più solamente militari impone, quindi, a tutti noi un approfondimento del concetto di sicurezza, cioè l'analisi specifica di nuove strategie geopolitiche. Ormai la politica si intreccia con l'economia, la cultura con le nuove tendenze tecnologiche, la sicurezza con le accresciute possibilità di comunicazione. È la dimostrazione che la globalizzazione ha ampliato fortemente gli orizzonti e gli scopi della politica per la sicurezza, ora più che mai urgenti e indispensabili. Non di meno, sono lodevoli le disposizioni con cui si stabiliscono in maniera chiara le modalità di finanziare gli interventi e con cui si stabiliscono i trattamenti economici, gli *status* giuridici, i trattamenti previdenziali e quanto ne consegue, per il personale sia militare che civile. In conclusione, signor Presidente, più volte viene ricordato come la nostra partecipazione alle missioni sia un modello sia dal punto di vista umano che militare: è con questo spirito e con questi auspici che noi del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE

siamo di fronte ad un provvedimento che aveva come obiettivo il superamento della prassi delle emergenzialità nel delicatissimo campo delle missioni internazionali. Oggi il nostro Paese partecipa a 24 missioni e nel corso degli anni abbiamo partecipato ad oltre 120 missioni. E siamo alla vigilia di un intervento militare in Libia, come ha confermato il ministro Pinotti solo poche settimane fa. La formulazione definitiva della legge non ci convince. Troviamo il testo un compromesso evidente, ma insufficiente, su una serie di punti: il processo autorizzatorio, la tipologia di missioni cui l'Italia può partecipare e, non ultimo, il ruolo di controllo del Parlamento. Avevamo presentato a maggio del 2013 una proposta di legge per regolamentare le missioni internazionali, prevedere l'indicazione puntuale delle fonti primarie al fine di restringere gli ambiti di intervento delle operazioni e delle missioni con l'obiettivo di garantire un più incisivo controllo del Parlamento. Questo è necessario perché sul piano internazionale si è affermata nel tempo una prassi caratterizzata da gravi violazioni ed ambiguità, e il nostro Paese ha partecipato a missioni ad alto contenuto di uso della forza, ed ha preso parte, anche con propri mezzi, ad operazioni di bombardamento. Abbiamo inoltre partecipato a missioni in cui mancava l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza ONU per azioni coercitive da parte di un'organizzazione o di un accordo regionale che invece è previsto essere esplicita e preventiva. Il testo oggi in discussione e la formulazione dell'articolo 1 a nostro giudizio non sono purtroppo sufficienti a dare forza al nuovo diritto internazionale, che riconosce la pace quale diritto fondamentale delle persone e dei popoli. Sarebbe stato importante indicare la tipologia delle missioni: non è pleonastico rispetto al riferimento alla legalità internazionale, ma al contrario la loro indicazione metterebbe al sicuro anche nel caso di eventuali operazioni NATO, perché - come sappiamo - anche la NATO deve comunque agire secondo la Carta delle Nazioni Unite e così non è sempre avvenuto. Per la procedura di autorizzazione delle missioni internazionali abbiamo sostenuto la necessità di superare la prassi che si è sviluppata negli anni e che ha limitato il ruolo del Parlamento alla sola autorizzazione dell'erogazione dei mezzi finanziari, non consentendo la possibilità di valutare compiutamente la coerenza delle missioni con il dettato costituzionale dell'articolo 11 e mettendo tutte le missioni sullo stesso piano. di legge non risponde alla necessità di maggiore coinvolgimento del Parlamento: l'articolo 2 lascia in capo al Governo la deliberazione della partecipazione alle missioni internazionali e solo successivamente prevede il passaggio alle Camere per la loro Il 25 febbraio scorso si è riunito il Consiglio supremo di difesa, analizzando anche la missione militare in Libia, con la ministra Pinotti che ha di fatto annunciato l'intervento, specificando che un intervento militare di occupazione è assurdo. Bene, allora di che intervento parliamo?

che introduce l'adozione di misure di*intelligence* di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenze all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale. Ricapitolando, si tratta del famoso emendamento Latorre, Il 15 settembre l'atto arriva in discussione in Aula al Senato, ma la discussione del disegno di legge quadro viene via via rinviata. Il 30 ottobre il Governo emana il decreto-legge n. 174 di proroga delle missioni internazionali; il testo viene definitivamente approvato dal Senato il 3 dicembre e, nel corso dell'esame, viene introdotto il famoso articolo 7-*bis* fotocopia dell'emendamento Latorre, rispetto avevamo presentato un emendamento soppressivo, cogliendo la pericolosità di quella norma. Questo articolo può essere utilizzato infatti alla prima occasione per dimostrare che si possono utilizzare militari in Libia

su richiesta delle autorità libiche, i corpi militari speciali italiani potranno entrare in azione grazie ad una legge approvata lo scorso novembre dal Parlamento, che permette ai gruppi di *élite* di agire seguendo la catena di comando dei servizi segreti. Il Governo, dunque, ha pervicacemente utilizzato il decreto di rifinanziamento delle missioni per aggirare il voto del Parlamento sull'intervento militare in Libia ed evitare la discussione su questo disegno di legge. Ma i cittadini italiani - ne siamo convinti - hanno diritto di conoscere sapere se l'Italia sta entrando in guerra con i suoi militari; sarà questo l'oggetto della discussione che faremo tra poco con il ministro Gentiloni. Ma noi chiediamo, in maniera particolare alla ministra Pinotti,

a proposito dei *raid* USA che sono partiti e che hanno già prodotto tantissime vittime civili, oltre che tra i miliziani jihadisti. Persino il «Wall Street Journal», una settimana fa, ha scritto che l'Italia si era rifiutata di permettere analoghi *raid* per paura di sollevare enormi polemiche interne ed alimentare nell'opinione pubblica un'opposizione contro la guerra, soprattutto se dovessero esserci vittime civili. costituisce per noi una preoccupazione gravissima e seria, anche perché la ministra Pinotti ha affermato più volte che, nel passato, accelerazioni unilaterali non hanno aiutato la Libia ad avere un futuro armonico. Vi state quindi contraddicendo continuamente e state prendendo in giro la Costituzione, la Carta delle Nazioni Unite e il popolo italiano. Tutto questo conferma soltanto che il Parlamento, sulla base di questo provvedimento, non avrà funzioni di controllo. Il testo unificato prevede una sessione parlamentare attraverso la presentazione di una relazione del Governo, ma noi abbiamo sostenuto la necessità di istituire un Comitato parlamentare di controllo che potesse avere Il testo si limita invece a fotografare l'esistente, scegliendo di non innovare come sarebbe stato Questo per noi è rilevante ed attuale, perché discutere della rispondenza delle missioni è un obiettivo fondamentale. Alcune scelte politiche, militari, geopolitiche e geostrategiche fatte nel corso degli ultimi anni si sono rivelate sbagliate e, anzi, completamente fallimentari

è stata persa l'occasione di presentare in sede internazionale una legge per riconoscere l'impegno del nostro Paese a promuovere il nuovo diritto internazionale, che ripudia la guerra e disciplina l'uso della forza come elementi di sovranazionalità e per finalità diverse da quelle belliche. Abbiamo perso l'occasione di smilitarizzare il profilo della nostra politica estera e scongiurare la possibilità che l'Italia si ritrovi a partecipare a missioni di guerra, così come avvenuto negli scorsi anni.

la partecipazione ad azioni ed interventi di guerra o l'uso della violenza bellica non devono essere più delegati ad organismi internazionali come la NATO, aggirando l'articolo 11 della Costituzione. priorità politica del nostro Paese gli interventi di carattere umanitario e non bellico, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto alla pace di ogni individuo e popolo, a cominciare dalle gestioni di crisi aperte

fornire una cornice normativa unitaria per l'invio di contingenti italiani all'estero, nel quadro delle missioni dell'ONU e delle altre organizzazioni cui partecipa l'Italia (in primo piano, la NATO e l'Unione europea). scenari di guerra ventilati per l'attuale situazione libica e l'eventuale intervento italiano nel Paese nordafricano rendono ancor più necessaria una legge che dia al Parlamento un ruolo chiave per la discussione e l'autorizzazione di eventuali iniziative militari,

era ampiamente condivisa da tempo e riconosciuta da tutti. Infatti, la Costituzione italiana non contiene previsioni che disciplinano l'impiego dello strumento militare all'estero, ad eccezione delle disposizioni sullo stato di guerra. Neppure esistono riferimenti normativi organici, al di là di alcune previsioni di principio contenute nella legge sull'ordinamento delle Forze armate, così come non esiste una normativa di carattere generale che disciplini i profili concernenti il trattamento economico e normativo il quadro giuridico per la partecipazione alle missioni viene definito essenzialmente con lo strumento del decreto-legge, che puntualmente il Governo sottopone all'approvazione del Parlamento Questo comporta una provvisorietà e disorganicità delle disposizioni e una grande precarietà delle stesse, soprattutto dal punto di vista finanziario, Il disegno di legge copre tutte le tipologie di missioni che si sono progressivamente andate definendo nel corso degli ultimi anni, da quelle di mantenimento della pace a quelle di conseguimento della pace, fino agli interventi umanitari, fornendo una serie di strumenti per una migliore programmazione degli stessi. ascoltando il suo suggerimento, mi avvio alla conclusione. Al di là del contenuto e delle altre disposizioni contenute nel provvedimento, bisogna sottolineare come il disegno di legge d'iniziativa parlamentare sia stato approvato alla Camera dei deputati senza alcun voto contrario. Tutto ciò è a conferma del fatto che l'esigenza di un nuovo intervento in questo settore fosse avvertito da tutti, maggioranza e minoranza.

quelle di cui si occupa questo disegno di legge. Vado a leggere testualmente il paragrafo 35: «Scarsità di risorse naturali. Le Nazioni in via di sviluppo hanno bisogno di crescenti livelli di energia e di materie prime per sostenere la loro crescita. La competizione per tali risorse potrebbe produrre un più elevato livello di tensione internazionale con conseguenti possibili conflitti. Più grave è la crescente scarsità di risorse vitali, quali l'acqua e il cibo, generata dalla crescita demografica, dai mutamenti climatici e da un utilizzo irrazionale dei territori. Essa è alla base di fenomeni di migrazione e potrebbe portare a una forte competizione, anche armata, per il possesso di tali risorse». Non è solo questa ipotesi appena letta a preoccuparci. In realtà, ve ne sono altre e vorrei illustrarvi un altro passaggio, sempre tratto dal Libro bianco. paragrafo 211 «Le Forze armate del prossimo ventennio saranno caratterizzate da un modello di tipo professionale, da dimensioni limitate e dall'esigenza di operare, sovente lontano dalla Patria o dalle basi di stazionamento, in ambienti conflittuali e complessi. L'esigenza è, pertanto, quella di un insieme di forze giovani, numericamente flessibile, professionalmente ben preparato e con una struttura del personale snella e ben proporzionata tra gradi, ruoli e specialità. Questo complesso di forze, inoltre, dovrà avere un elevato grado di "utilizzabilità operativa", essere cioè idoneo a operare in ambienti difficili, lontani dalle sedi stanziali anche per lunghi periodi e quindi in grado di accettare minori vincoli di natura extra-professionale, essere fisicamente idoneo e predisposto al sacrificio personale». Questo è il mondo che immaginate e che state preparando ai nostri giovani. Noi immaginiamo un futuro differente, in cui ci si prepari davvero alla pace, iniziando a riconvertire le nostre fabbriche di tecnologia bellica, creando un'industria supportata da adeguata ricerca e sviluppo, tesa alla realizzazione di prodotti per il benessere delle persone, per tecnologie che ci permettano di creare quell'autosufficienza energetica o che vi tendano oppure per un'agricoltura che copra il nostro fabbisogno alimentare e allo sfruttamento delle immense ricchezze culturali, storiche e paesaggistiche del nostro bellissimo territorio. Apro una parentesi riguardo a quanto appena detto. L'amico e collega Cioffi mi faceva notare l'altro giorno che la Germania, ad esempio, ha prima creato l'industria del fotovoltaico e poi ha fatto una politica di incentivi agli impianti per i cittadini, i quali hanno comprato i prodotti tedeschi. L'Italia invece, in leggera controtendenza, ha incentivato prima il fotovoltaico e gli italiani ovviamente hanno acquistato prodotti tedeschi. Tornando a noi, mi si potrà obiettare che il nostro Paese non ha materie prime e che per esse dipendiamo dal resto del pianeta. Per questo dobbiamo proteggere gli approvvigionamenti energetici, i nostri commerci e le vie di comunicazione verso i mercati, dato che siamo un'economia di trasformazione. Qui arriviamo a un'altro punto dolente: non solo avete una pessima visione del futuro, ma avete - perdonatemi - anche una cattiva gestione del presente. Non ritenete corretto informare il popolo italiano su quali siano le reali motivazioni delle missioni internazionali? Non pensate sia giusto che i cittadini sappiano che i nostri soldati andranno in guerra, forse in Libia, affinché noi si possa godere del gas libico? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non sarebbe il caso di dire chiaramente, volta per volta, quali siano gli interessi nazionali reali? Sarebbe opportuno fare esprimere gli italiani su questi temi. Se proprio non lo si vuole, almeno si faccia decidere il Parlamento. Invece voi no; volete che a decidere sia solo il Primo Ministro e ne siete pure orgogliosi. Lo avete messo nero su bianco: il Parlamento non può nemmeno negare l'autorizzazione. Riteniamo doveroso informare e discutere senza ipocrisia quali siano gli obiettivi di ogni singolo utilizzo delle nostre Forze armate o di sicurezza. Abbiate il coraggio di dire che, se si vuole mettere benzina nell'automobile, è possibile che ci siano dei morti, magari non italiani, magari nigeriani o iracheni. Mi sia consentito di utilizzare parole di altri: il desiderio di mantenere la pace o esportare la democrazia è stato storicamente utilizzato come artificio retorico per giustificare ogni tipo di aggressione armata. Raramente un invasore ha mosso un attacco senza proclamare a gran voce il suo intento pacificatore. Volete dire agli italiani che alcune missioni servono o serviranno esclusivamente per potersi ingraziare le potenze straniere? Per il prestigio, per poter valere sul piano internazionale ai tavoli ONU e NATO (che secondo noi sarebbero organismi da modificare)? Credo che sia ora di porre fine al tempo del «Ce lo chiede l'Europa», «Ce lo chiede la NATO» o «Ce lo chiede l'ONU». Fare un piano serio per il futuro, fissando chiaramente quali sono le priorità dell'Italia, non significa rinnegare i trattati o mancare di lealtà; significa semplicemente pensare un mondo diverso e magari sarà questo un modo per convincere altre Nazioni a farlo. Un'ultima nota: a breve arriverà l'ennesimo decreto-legge sulle missioni e saremo impegnati nuovamente su questi temi. Stessa farsa di sempre: urgenza, urgenza, urgenza. Questo disegno di legge poteva essere approvato già da molto tempo. Non so se lo volete veramente approvare. Presidente, termino dichiarando il voto di astensione del nostro Gruppo, sapendo che una legge che disciplini le missioni internazionali sia realmente necessaria. Abbiamo provato a migliorarla, abbiamo dato il nostro contributo abbiamo cercato di dare centralità al potere decisionale del Parlamento, ma non avete voluto ascoltarci. Ora approvatevela. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione finale di questo importante disegno di legge arriva in un momento particolare che vedrà il nostro Paese impegnato in prima linea sulla crisi libica. Arriva, tale discussione, nei giorni della liberazione di due nostri connazionali sequestrati in Libia, una gioia che non mitiga, però, la profonda amarezza per la perdita degli altri due e non attenua le ombre che hanno accompagnato questi eventi. Spiace inoltre registrare la nota stonata del *Premier* che, pur trovando cinquanta minuti del suo prezioso tempo per accomodarsi in un benevolo salotto televisivo domenicale, non ne avrebbe trovato uno per comunicare la gentilezza del cordoglio ai familiari dei connazionali trucidati, né allevia che il Ministro degli affari esteri abbia avvertito tale sensibilità dopo qualche giorno dai tragici eventi. Detto ciò, comprendiamo come vi sia la necessità, in questo delicato frangente geopolitico, di costruire anche in Parlamento un clima che dia ai nostri militari, una volta di più, la giusta percezione di un Paese unito, ove mai venissero impiegati in una missione internazionale a guida italiana. D'altra parte, è lecito pensare a tale evenienza poiché, se da un lato risultano apprezzabili i tentativi di pervenire in Libia al miraggio di un governo unitario, bisogna mettere in conto che si potrebbe arrivare ad esiti non più diplomatici, poiché più cresce l'instabilità, più si rafforza l'ISIS. In tale scenario, assistiamo da tempo ad una spasmodica voglia del nostro Governo di assunzione della responsabilità di comando dell'eventuale coalizione, gridando ai quattro venti questa smania, col rischio di rendere il Paese più esposto alle ritorsioni. Certo, siamo geograficamente i più vicini a quel Paese, dobbiamo tutelare i nostri confini dal rischio terrorismo e i nostri preponderanti interessi energetici in Libia. Libia. Quella del Governo italiano sembra però una brama di comando, quasi come un tentativo di riscatto da una politica estera deficitaria e balbettante, appaltata per lo più agli alleati, essendo divenuto il nostro Paese quasi una sorta di collaboratore familiare degli Stati Uniti, i quali decidono per noi se dobbiamo rimanere in Afghanistan, se dobbiamo inviare più soldati in Iraq, se dobbiamo concedere loro la base di Sigonella. Li abbiamo assecondati in più occasioni, anche su scelte che sembravano già al tempo scellerate, dalla guerra in Iraq a quella disgraziata in Libia. Pazienza se, nel frattempo, intercettavano il nostro Presidente del Consiglio e ancora oggi, a qualche settimana dalla scoperta, non risultano scuse ufficiali, col Governo italiano che si limita a docili parole di circostanza. Forse, però, signor Presidente, ci permetteranno di guidare la missione in Libia, di aiuto e di stabilizzazione di quel Paese, di cui tanto si parla. Molte grazie, vorremmo capire meglio quale sarà il contributo di quei Paesi, che in realtà sono i principali responsabili dell'attuale disastro libico. La guerra in Libia l'hanno voluta, innanzitutto, i francesi e i britannici e ha portato solo disastri e caos, di cui noi piangiamo più di altri le conseguenze. Prima di imbarcarci in pericolose avventure, si valuti allora con estrema attenzione ciò che, pur apparendo un doveroso omaggio al prestigio, ai legami storici dell'Italia col «bel suol d'amor», potrebbe in realtà essere una polpetta avvelenata. Prima di avanzare richieste di comando, sarebbe opportuno capire quale sarà la quota in termini di uomini e mezzi di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, di quei Paesi che, nel 2011, assunsero la pessima decisione, subita dall'Italia, anche per le pressioni interne ai più alti livelli, di intervenire in Libia, trasformando di fatto quel Paese in uno Stato fallito. Oggi la Libia costituisce una seria minaccia per l'intera area del Mediterraneo a causa di quelle sciagurate valutazioni e dell'avallo alle rinomate primavere arabe che condussero i *leader* occidentali, il presidente Obama in testa, ad allearsi in Egitto con i Fratelli musulmani e in Siria a sponsorizzare, finanziare ed armare i cosiddetti ribelli anti-Assad, tra cui si annidavano anche gli invasati che vogliono distruggere la nostra civiltà. A questi Paesi nostri alleati spetterebbe, in primo luogo, porre rimedio alla vicenda libica, al netto del prestigio che deriverebbe all'Italia, ove dovesse mai assumere la guida della coalizione internazionale, confermatale per ora solo a parole. Vorremmo poi capire, nel caso di eventi bellici e di comando italiano delle operazioni, cosa verrà riservato a quelle regioni, che per questioni geografiche dovessero trovarsi in prima linea, mentre si avvicina la stagione turistica. Sono stati per caso studiati, signor Ministro, oltre i piani bellici, eventuali benefici e compensazioni per questi territori? Ad ogni modo, la stessa frenesia nel richiedere il comando delle operazioni non l'abbiamo ravvisata per stroncare il traffico di migranti, col suo carico di disperazione e di vittime. Il Governo ha seguitato a cavalcare le onde emotive che hanno finito per stancare l'opinione pubblica italiana, incalzata dal rischio terrorismo e da un'immigrazione incontrollata. Ci aspettiamo che, non appena sarà deciso l'eventuale intervento, col benestare delle autorità libiche, non una sola barca dovrà salpare da quei porti e che i centri di accoglienza vengano creati lungo le coste libiche. La mancanza di energia del Governo italiano nell'affrontare sino ad oggi seriamente il problema è stata ad un passo dalla complicità con i trafficanti di uomini. Dovete fugare questi dubbi, che qualcuno, cioè, all'interno del Governo - non certo il ministro Pinotti - abbia interesse a mantenere questo baraccone, per il criminale cinismo di quanti dal fenomeno migratorio traggono benefici economici e politici. Per tornare all'argomento in discussione, Presidente, il nostro Gruppo esprimerà un giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge in esame, che supera l'attuale disciplina incentrata sulla decretazione d'urgenza, una modalità desueta, con cui le Camere si esprimevano con un provvedimento quasi sempre a ridosso della scadenza dei decreti. Con tali norme viene definito un quadro caratterizzato da certezze giuridiche e garanzie funzionali, oltre che da certe coperture economiche delle missioni internazionali cui parteciperà il nostro Paese. Il testo è arrivato in Senato dopo la prima lettura della Camera, ove Forza Italia ha già dato un importante contributo al varo di una legge attesa da molte legislature. il nostro Gruppo voterà a favore per il particolare riguardo che da sempre ripone verso le Forze armate, soprattutto quando i nostri militari, a tutela dei quali il disegno di legge in esame viene varato, svolgono impegnative e delicate missioni all'estero. È utile ricordare che le missioni militari rappresentano un punto qualificante della nostra politica estera, tanto più in un tempo di grave e pericoloso deterioramento della sicurezza in Medio Oriente e nel Nord Africa, con una seria minaccia alle porte di casa. Il disegno di legge in argomento garantisce che l'uso della forza militare si realizzi sempre nel rispetto della Costituzione e nel quadro degli organismi e degli impegni internazionali, dal nostro Paese mai disattesi, con uno zelo a volte eccessivo che andrebbe, invece, praticato con più oculatezza, in modo più rispondente ai nostri interessi strategici. Ciò anche in virtù dei continui tagli al bilancio della difesa, colpevolmente ridotto ormai quasi all'1 per proprio quando più seria si fa la minaccia del terrorismo agli equilibri internazionali. Ad ogni modo, con la previsione di un fondo annualmente inserito nella legge di stabilità, sarà consentito alle Camere di esprimere un giudizio su ciascuna missione

per la politica estera e di difesa del nostro Paese. In ultimo, signor Presidente, oggi è accaduto un fatto di assoluta rilevanza per cui bisogna dare atto alla sperimentata sensibilità del Presidente della Commissione difesa, il senatore Nicola Latorre *(Applausi dei in questo ramo del Parlamento, a quell'inconcepibile forzatura per la quale la maggiore forza parlamentare di opposizione era tenuta fuori dall'organismo parlamentare di controllo dei servizi segreti; una questione stancamente protrattasi, differita e rinviata, non più tollerabile, soprattutto nel momento in cui agli apparati di *intelligence* sono state attribuite nuove, giuste ed importanti funzioni. Tale risultato, oltre per l'impegno del senatore Latorre, è stato reso possibile anche in virtù dell'attività e dello scrupolo coscienzioso profusi dal Presidente del Senato, che ringraziamo per quanto fatto. Ci auguriamo, pertanto, che la Camera dei deputati provveda quanto prima a ratificare l'importante disegno di legge

Sono passate ben quattro legislature con diversi tentativi, ma mai si era riusciti a trovare una soluzione che mettesse d'accordo Governo e Parlamento. In primo luogo, il mio ringraziamento per il prezioso lavoro svolto va ai relatori, al Governo che ha facilitato il lavoro e contribuito alla definizione di una sintesi che ci consente di arrivare ad un risultato tanto atteso; va anche a tutti i colleghi delle Commissioni affari esteri e difesa per i miglioramenti che sono stati introdotti nel provvedimento. Il disegno di legge che il Senato si accinge ad approvare non è di quelli che troviamo sulle prime pagine dei giornali e che occupano i dibattiti, ma costituisce senza dubbio un punto di avanzamento per il nostro ordinamento e per la politica estera e di difesa del nostro Paese; ciò nella consapevolezza che il quadro delle missioni è mutato radicalmente e progressivamente negli ultimi anni, con ripercussioni già oggi presenti e che si avranno ancora inevitabilmente di più sulla politica delle difesa e sulla politica estera. Valenza ed effetti di questo provvedimento sono profondi e importanti: in primo luogo, come è stato osservato da molti nel dibattito parlamentare, viene finalmente introdotto un quadro normativo che attribuisce maggiore certezza e coerenza alla nostra partecipazione alle missioni internazionali, facilitando un maggiore approfondimento da parte del Parlamento sulla risposta necessaria per affrontare crisi complesse come quelle di oggi e una migliore e più proficua interazione sul tema fra le distinte prerogative del Presidente della Repubblica, del Governo e delle Camere. In questo senso sta il punto fondamentale e, se vogliamo, di novità rispetto ai tentativi infruttiferi del passato e che riguarda il tanto discusso processo autorizzativo delle missioni. Un aspetto cruciale, in cui si è trovata una convergenza ed un punto di equilibrio tra poteri e prerogative garantite dalla Costituzione al Parlamento ed al Governo. Ma la rilevanza del testo sta soprattutto nell'esprimere le linee di azione e cultura politica che rappresentano una opzione irrinunciabile per l'Italia, i principi base che orientano e sovrintendono alla nostra politica estera e di sicurezza, principi che seguiamo da molti anni e discendono dal secondo periodo dell'articolo 11 della nostra Costituzione e che oggi vengono esplicitati in un testo normativo. Mi riferisco alla nostra adesione al sistema di relazioni e istituzioni basato sulle Nazioni Unite e le altre organizzazioni cui apparteniamo in conformità al diritto internazionale, e quindi alla nostra scelta per la gestione multilaterale delle crisi e per conferire stabilità, continuità e capacità di programmazione all'azione della comunità internazionale a favore della stabilità e dello sviluppo pacifico. Le missioni internazionali rappresentano un'assunzione di responsabilità per un Paese come il nostro, che si è sempre schierato dalla parte della tutela del diritto internazionale e vanta un impegno di lunghissimo periodo a favore dei diritti umani, per la gestione multilaterale delle crisi e per il rafforzamento delle organizzazioni multilaterali in uno scenario mondiale sempre più esposto a rischi di conflitto, dove, tra l'altro, possiamo ben dire che, se vogliamo essere fruitori di sicurezza nell'interesse del nostro Paese, dobbiamo con coraggio e, appunto, responsabilità, essere contemporaneamente produttori di sicurezza. Colleghi, poco più di un anno fa, il 1° agosto 2014, questa stessa Assemblea ha approvato in via definitiva la riforma della cooperazione internazionale per lo sviluppo. Anche di quella riforma non si è parlato molto e anche questa, invece, è un riforma estremamente rilevante, che articola e definisce l'impegno del nostro Paese a incidere sulle cause più profonde dei conflitti e a favore della stabilità tramite l'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui. Parimenti, i decreti attuativi della legge n. 244 del 2012 di riforma dello strumento militare e la definizione del Libro Bianco della difesa, con le successive determinazioni che il Parlamento dovrà assumere, possono essere considerate una vera riforma di sistema e testimoniano la centralità, sul piano strategico, che le Forze armate rappresentano nell'agenda politica. Credo che questi provvedimenti nobilitino il lavoro di Governo e Parlamento in questa legislatura e diano il segno del lavoro che viene compiuto di riforma ed evoluzione del nostro ordinamento. Colleghi, questa fase storica vede un arco di crisi estremamente complesse e la nostra politica estera deve sapere cambiare e adeguarsi, fungendo anche da stimolo alle altre democrazie. Partecipare alle missioni internazionali è in primo luogo, come detto, un atto di responsabilità; in secondo luogo, esserci ed esprimere un contributo, tra l'altro di notevole livello, offre all'Italia uno spazio politico di rilievo per poter incidere nei percorsi di decisione. È in tale contesto che il nostro Paese è riuscito, con la missione *Mare nostrum*, a inserire nell'agenda dell'Unione europea la questione del Mediterraneo, che oggi ha portato a EUNAVFOR MED, e la questione libica, su cui il nostro Governo si sta adoperando affinché le condizioni politiche consentano finalmente il varo definitivo di un Governo solido e pienamente legittimato di unità nazionale, proprio perché si ha la consapevolezza che l'efficacia di un intervento di stabilizzazione dipenda dal presupposto politico. con l'autorevolezza dell'intervento del ministro Gentiloni, non c'è dubbio che siano indispensabili una strategia politica concreta e un progetto di stabilizzazione che deve rientrare

voglio ricordare che il nostro Paese, con l'unica eccezione della missione in Iraq del 2003, si è sempre mosso in piena aderenza al diritto internazionale e quindi nell'ambito di missioni autorizzate dalle Nazioni Unite. Un'eventuale nostra partecipazione ad un impegno internazionale non potrà che avvenire con questi presupposti e con i necessari passaggi istituzionali. Basta guardare a quanto avvenuto, ad esempio, per il nostro sostegno all'impegno contro il Daesh in Iraq, e all'interlocuzione tra Governo e Parlamento che abbiamo seguito, e non può non constatarsi che questa è la nostra prassi. Ora, non c'è dubbio che il Mediterraneo e la Libia rappresentino una priorità assoluta per il nostro Paese. E non c'è dubbio che la minaccia jihadista in Libia (la crescita del Daesh, la presenza di gruppi salafiti che si rifanno ad al-Qaeda come Ansar al-Sharia a Bengasi e a Derna, e la possibile entrata in scena di altri gruppi jihadisti

ma siamo e resteremo saldamente incardinati all'interno delle organizzazioni che da decenni sono i nostri ambiti di riferimento. L'argomento delle missioni internazionali, quindi, è tra i più delicati, chiamando in causa temi sensibili come la libertà e la vita umana, che richiedono un altissimo senso di responsabilità. Le Forze armate sono diventate strumenti funzionali alla sicurezza ed alla stabilità internazionale e desidero ulteriormente ricordare che tutte le missioni internazionali dell'Italia hanno ottenuto riconoscimenti unanimi dalle autorità sia politiche che militari dei Paesi in cui hanno operato inoltre, i nostri militari hanno saputo sempre entrare in sintonia con le popolazioni stanziate nei vari teatri in cui si sono trovati ad intervenire. In conclusione, voglio esprimere gratitudine ai nostri militari, senza dimenticare il tributo offerto, anche e sopratutto in termini di vite umane, dai nostri soldati, che è stato altissimo e che ha testimoniato, anche sotto questo aspetto, il valore di eccellenza che da sempre contraddistingue la nostra presenza nel contesto delle missioni internazionali. contesto delle missioni internazionali. Il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento, che consideriamo una vera e propria riforma, in cui si rafforza un'intesa tra Governo e Parlamento e che ci porterà lontano, perché pensiamo che a conclusione dell'*iter* parlamentare, con questa legge, il nostro Paese sarà più forte e il Partito Democratico, ancora una volta, con orgoglio e volontà, è per la piena collocazione internazionale dell'Italia, per il diritto internazionale e la stabilità, nella consapevolezza che questa impostazione consente all'Italia quella capacità internazionale indispensabile per affrontare questioni complesse nello scenario globale.

di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Gentiloni Silveri.

Signor Presidente, onorevoli senatori, l'informativa del Governo sulle scelte relazione alla crisi libica si intreccia, come sappiamo tutti, con la drammatica vicenda dei nostri connazionali sequestrati

Non possiamo che iniziare questa informativa, quindi, con un messaggio comune di cordoglio e vicinanza alle famiglie. All'inizio della mia informativa riferirò sugli elementi che abbiamo a disposizione, fermo restando che, dopo le prime informazioni che sono già state rese dal sottosegretario Minniti, il Copasir sarà aggiornato continuamente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane degli sviluppi

che è una *joint venture* tra ENI e la National oil corporation libica. In quel momento, un gruppo di quattro connazionali composto da Salvatore Failla, Filippo Calcagno, Fausto Piano Gino Pollicardo, impiegati presso la ditta Bonatti, provenienti a bordo di un minivan dal confine libico-tunisino di Ras Agedir, è stato raggiunto e fermato da due veicoli SUV. Dai SUV sono scesi uomini armati a volto coperto, alcuni dei quali avrebbero indossato uniformi di tipo militare. Questi hanno sequestrato i quattro cittadini italiani lasciando sul posto l'autista libico, che era originario di Sabrata e lavorava da circa un anno per la ditta Bonatti. Non sono emersi elementi di riconducibilità a formazioni di Daesh in Libia. Non è mai giunta alcuna rivendicazione. Tra le principali ipotesi in corso, la più accreditata è quella di un gruppo criminale filoislamico operante tra Mellitah, Zuara e Sabrata. L'*intelligence* italiana ha tempestivamente attivato tutte le risorse disponibili, umane e tecnologiche, e ovviamente ogni collaborazione possibile con i *partner* della regione e internazionali, per il coordinamento a livello centrale e la cooperazione in ambito periferico. Costante è stato il rapporto tra *intelligence* e Unità di crisi della Farnesina. Nell'ambito dell'attività condotta dall'*intelligence* sono state acquisite informative da fonti umane e approfondimenti di natura tecnica, senza però mai riuscire a localizzare con sicurezza e precisione i possibili luoghi di detenzione. Nel pomeriggio del 2 marzo, nell'ambito di quotidiane azioni di controllo del territorio condotte dalle forze locali facenti capo alla municipalità di Sabrata, un convoglio composto da due o tre *pickup* (del tipo Toyota Tundra), nell'area a Sud di Sorman, è stato ingaggiato in un conflitto a fuoco che ha provocato nove vittime, tra cui purtroppo i nostri due connazionali, che erano stati prelevati dal nascondiglio dove erano detenuti insieme agli altri due colleghi italiani, probabilmente allo scopo di spostarli in due movimenti differenti. Nelle prime ore del mattino del 4 marzo, Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, lasciati incustoditi nel luogo di prigionia, sono riusciti a fuggire e a raggiungere la municipalità di Sabrata, mettendosi in contatto con le famiglie e con le autorità tripoline e italiane. Sulla base delle evidenze emerse, i quattro connazionali sono stati nelle mani dello stesso gruppo durante tutta la durata del sequestro, cambiando, prima degli eventi citati, solo una volta il luogo di prigionia. Per proprie finalità, il gruppo dei sequestratori ha lasciato intendere che gli ostaggi fossero stati separati o passati di mano ad altri gruppi, fatto che in questi ultimi giorni si è rivelato non essere vero. Voglio infine chiarire che non è stato pagato alcun riscatto, che non risulta fosse imminente la liberazione degli ostaggi e che non risulta siano stati trovati nel nascondiglio passaporti appartenenti ad elementi di Daesh. Lo dico, onorevoli senatori, perché la ricerca della verità è doverosa, vede impegnata la procura di Roma e il Parlamento giustamente la esige, ma questo non vuol dire in alcun modo avallare voci e insinuazioni che provengono da un contesto interessato ad ogni forma di strumentalizzazione. È in circostanze come queste, onorevoli senatori, che il Parlamento è chiamato a mostrare il volto di un'Italia coesa, che si stringe attorno alle famiglie delle vittime, che saluta i connazionali che si sono salvati, che si unisce agli apparati di sicurezza impegnati sul campo, ancora in queste ore, per il rientro delle salme. Un grande Paese si comporta così, almeno in questi casi, lasciandosi alle spalle *bagarre* e contrapposizioni di parte. Il sequestro e perfino le modalità penose del rientro dei nostri connazionali ripropongono alla nostra attenzione la criticità e la pericolosità della situazione in Libia. A cinque anni dalla caduta di Gheddafi, il Paese è diviso, frammentato, attraversato da un'alta conflittualità vede una presenza di Daesh e di diverse formazioni jihadiste. Di fronte a questo quadro, credo che il Parlamento debba innanzitutto interrogarsi partendo dal nostro interesse nazionale. Qual è il nostro interesse nazionale? Il nostro interesse nazionale è quello di evitare che il processo di disgregazione in atto prosegua o addirittura si accentui. Evitare il collasso della Libia, insomma; evitare un collasso che trasformerebbe quel Paese in una polveriera, oltre ad accentuare una già incipiente crisi umanitaria. Gli «Stati falliti» sono ormai più pericolosi degli «Stati canaglia», ha detto il presidente Obama all'ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Evitare il collasso, dunque, e ritessere la tela della sovranità. Serve un Governo legittimo, capace di riconciliare Tripolitania, Cirenaica, Fezzan l'enorme quantità di milizie presenti in Libia, di riacquisire gradualmente - non sarà un'operazione di poche settimane - il controllo del territorio, di prosciugare l'acqua nella quale nuota Daesh, di contrastare il traffico di essere umani, da cui derivano i flussi di immigrazione clandestina, e di valorizzare le risorse libiche, che certamente non mancano. L'obiettivo di questo Governo, di un Governo capace di avviare questo percorso, è emerso a metà dicembre dalla Conferenza organizzata a Roma dall'Italia e dagli Stati Uniti, che ha reso possibile poi, sempre a dicembre, gli accordi di Skhirat in Marocco

Dal primo momento, non ho certo nascosto al Parlamento la fragilità del percorso avviato a Roma a metà dicembre. Del resto, come potrebbe non essere fragile un percorso nella regione di cui stiamo parlando, attraversata da un disordine permanente e drammatico? Come potrebbe non essere fragile in Libia? Chiunque conosca, anche da lontano, questo Paese, sa quanto complessa e frammentata sia quella realtà, non certo riconducibile soltanto alle due istituzioni

questa, onorevoli senatori, è la sola base su cui lavorare. C'è una maggioranza nell'organismo che, per così dire, deve dare la fiducia al nuovo Governo libico: mi riferisco alla maggioranza di 101

a New York le modalità per consentire a questa maggioranza, nonostante il boicottaggio degli estremisti, di esprimersi in qualche modo

caso, non facciamoci illusioni: sarà solo un primo passo. Poi, bisognerà includere altri settori e altre forze che oggi non partecipano a questo processo, perché il processo ha bisogno di maggiore inclusione e solidità.

a continuare a curare i feriti che si producono negli scontri in Libia. Il Governo legittimato farà le sue richieste ed è in questo scenario che lavorano, per la pianificazione, i Ministri della difesa, coordinati dal ministro Pinotti e dall'Italia. Lavoriamo per rispondere ad eventuali richieste di sicurezza del Governo libico, niente di più e niente di meno, nel rispetto della Costituzione visto che, come ho detto, c'è una risoluzione delle Nazioni Unite che lo prevede e, ovviamente, lo faremo soltanto in seguito al via libera da parte del Parlamento, come ha ricordato qualche giorno fa il Presidente del Consiglio. So bene che questo percorso ad ostacoli può apparire troppo lento. Vedo benissimo il consolidarsi di Daesh in Libia. Paradossalmente, è stato proprio il recupero del 40 per cento del territorio iracheno occupato da Daesh da parte della coalizione a spingere qualche elemento dei combattenti di Daesh verso la Libia. Oggi, secondo le nostre analisi, ci sono circa 5.000 combattenti di Daesh in Libia

Sul terreno, questi 5.000 combattenti sono contrastati spesso dalle milizie islamiche, soprattutto in Tripolitania. Sappiamo però che il pericolo di un macabro *franchising* di Daesh, cioè di gruppi locali che si uniscono al marchio del sedicente Stato islamico, è un rischio sempre presente. Da questa minaccia terroristica l'Italia deve difendersi e l'Italia si difenderà, come prevede l'articolo 52 della nostra Costituzione. Del resto, è questa la ragione per la quale il Parlamento a dicembre ha deciso che, in certi casi, operazioni d'*intelligence* possano richiedere condizioni di sicurezza assicurate dal supporto di unità militari e di tali operazioni il Parlamento sarà informato attraverso il Copasir, come prevede la legge n. 124 del 2007. Una cosa deve essere chiara: il contrasto al terrorismo deve basarsi su uno straordinario impegno informativo, quando necessario, su azioni circoscritte, su risposte proporzionate alla minaccia effettiva e concordate tra alleati. Tuttavia, non è dal contrasto al terrorismo che possiamo attenderci la stabilizzazione della Libia. Confondere legittima difesa con stabilità della Libia non aiuta; anzi, può provocare spirali pericolose. A chi agita la minaccia di Daesh, che è reale e dalla quale dobbiamo difenderci, per invocare interventi militari, rispondiamo che gli interventi militari non sono la soluzione; talvolta, possono perfino aggravare il problema. A chi snocciola cifre di soldati pronti a partire, magari perché gli italiani non possono sottrarsi perché così fan tutti, ricordo che la Libia è un Paese che ha un'estensione pari a sei volte quella e che ha circa 200.000 uomini armati, tra milizie ed eserciti di diversa bandiera. No, non è proprio un teatro facile per esibizioni muscolari. Insomma, il Governo non è sensibile al rullare di tamburi e non si farà influenzare da radiose giornate interventiste. Il Governo difenderà il Paese dalla minaccia terroristica con le azioni proporzionate che saranno necessarie. Il Governo interverrà, se e quando possibile, per rispondere alle richieste di sicurezza di un Governo legittimo e impegnato a riprendere gradualmente il controllo della sovranità del proprio territorio e lo farà su decisione del Parlamento e coordinando le forze alleate. Il Governo non si farà trascinare in avventure inutili e persino pericolose per la nostra sicurezza nazionale. Contiamo sul sostegno del Parlamento ad una linea che deve combinare fermezza, prudenza e responsabilità.

stiamo procedendo verso questa guerra in Libia che, ricordo, era il primo Paese, per sviluppo, del continente africano, con il 38 per cento di petrolio prodotto e l'11 per cento di *export* verso l'Europa.

panafricana. Da lì è partita tutta l'*escalation* che ci ha portato fino a qui, oggi. Lei identifica la Libia con l'ISIS, ma l'ISIS purtroppo molto spesso è un'entità che viene

da parte delle forze terroriste. Hanno una potenza militare irrilevante: sono il nulla che avanza nel niente, come sta affermando qualche analista. Probabilmente, credere che l'ISIS sia un pericolo sul piano militare, un pericolo così destabilizzante per l'Occidente, è come credere che un sindaco che non ha mai lavorato in vita sua possa scalare il primo partito d'Italia e diventare Presidente del Consiglio. Certo, se credete a questo, probabilmente crederete anche a quell'altro!

ad Ovest confina con gli Stati Uniti, è ovvio; a Sud-Ovest, invece, confina con cinque miliardi di investimenti italiani persi, 140 miliardi di reddito immediatamente dopo la guerra e 500 miliardi nel medio periodo; a Sud-Est, infine confina con circa tre miliardi annui di *export* di armi italiane, soltanto di armi italiane.

cinesi, francesi, britanniche e americane che stanno manovrando nel Mediterraneo non raccolgano i barconi degli immigrati, ma continuiamo a raccoglierli noi. Forse perché già è stato deciso - e voi vi state già predisponendo ad accertarlo in maniera supina - che Grecia e Italia gestiranno la crisi umanitaria. Concludo, Presidente,

ha dichiarato: vedo all'orizzonte il petrolio a 70-80 dollari al barile, ma serve la Libia unita. È questo il vostro grande miraggio! Ebbene, allora vi do un consiglio: preparatevi i vostri discorsi

salutiamo allievi, allieve e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Croce-Aleramo» di Roma, che seguono i nostri lavori. *(CoR)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, molto giustamente, a nostro avviso, l'onorevole Ministro ha voluto stamattina iniziare ricordando la drammatica vicenda dei nostri connazionali. Di fronte a quella drammatica vicenda, come parlamentari di opposizione ci onoriamo di dichiararci più che sensibili alle parole del Ministro quando invoca l'opposizione parlamentare

una legittima amarezza per i due connazionali che non ce l'hanno fatta e non ci vergogniamo di provare una legittima soddisfazione per i due connazionali che ce l'hanno fatta.

E riteniamo improprio che un Governo disposto ad adoperare, in sede politica e diplomatica, l'espressione «ricatto» a proposito di questa o quella vicenda politica, Erdogan, non usi tale espressione a proposito della restituzione delle salme dei due connazionali.

Ho trovato anche felice il suo richiamo a quell'immagine - mi pare del presidente Obama - per cui gli Stati falliti sono ormai più pericolosi degli Stati canaglia, e cioè

libiche, perché allora aspirava a un incarico dell'ONU che poi non ha avuto: è evidente che la Libia, come Stato,

affatto le sue valutazioni e la speranza italiana di uno Stato che si ricostituisca partendo dall'Esecutivo di uno Stato nazionale che ha bisogno di lasciar esprimere la maggioranza dei 101 deputati. Questa è un'espressione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e non solo dell'Italia, ma non è così. Non è il Governo il fattore dei fattori degli Stati. Preferirei che lei avesse usato un'espressione diversa: «lasciamo esprimere una maggioranza» e non «lasciamo esprimere un Parlamento o un segmento di Parlamento», poi aspirare che si possa arrivare ad un parlamentarismo libico, da Tobruk a Tripoli. È la sua immagine. Ma questo parlamentarismo, nella storia libica

sulla fragilità di un percorso che lei stesso ha definito tale, quello della Conferenza di Roma di metà dicembre, insieme agli americani, si sono sollecitate tante attese, tanti luoghi comuni e tante banalità, anche onusiane. Da questo punto di vista, l'atteggiamento dell'Italia è stato sempre di un lealismo ai limiti del servilismo nei confronti delle Nazioni Unite. stanno facendo sempre più errori in questa traiettoria di Stati falliti. Sulla passione per i beni numismatici del diplomatico spagnolo non voglio moralisticamente incrudelire, ma da parte delle Nazioni Unite ci sono soltanto riferimenti di banalità pacifistica

mai. Il problema - come ha detto con intelligenza il senatore Mauro - è la costruzione istituzionale del rapporto tra

che è stato in qualche modo certamente aggirato dalla procedura parlamentare e, se posso fare un processo alle intenzioni, dal terrore politico dei colleghi del PD di aprire la diatriba miserabile della costituzionalità della pace e della guerra, una storia francamente penosa che risale all'intervento americano in Iraq.

che io posso anche ritenere auspicabile, ma che non può andare a detrimento delle libertà degli altri parlamentari e dei modi di procedere nei lavori. Sono considerazioni che non riguardano lei, Ministro, che è stato colpito tangenzialmente dalla vicenda, ma semmai la Presidenza del Senato. Devo anche dire che in questo senso, a prescindere da quanto è avvenuto, non posso che apprezzare la sua espressione lessicale che a me, vecchio giolittiano, piace molto: questo non è un Governo da radiose giornate interventiste. Nella storia patria, le radiose giornate implicano il momento più laido dell'attacco al Parlamento, altro che il 1922. È una pagina oscura. Noi andammo in guerra senza passare per il Parlamento. L'antigiolittismo vide uniti personaggi a me cari: Albertini, il direttore del «Corriere della Sera», mandante degli squadristi di D'Annunzio; Einaudi e Salvemini. Fu sbagliatissimo e, quindi, ogni considerazione politica di prudenza è ben accetta. quello che non possiamo accettare è che nella politica estera italiana degli ultimi anni abbiamo visto due protagonismi esagerati. Uno è quello delle Nazioni Unite, sulla base di quanto dicevo prima, e l'altro - me lo consenta, senza il moralismo scandalistico del collega del Movimento 5 Stelle - è l'Ente nazionale idrocarburi, che alla Farnesina gioca un ruolo esagerato. La vicenda della visita del Presidente iraniano è stata, da questo punto di vista, maleodorante. E ci sarebbe anche piaciuto che in questa settimana - o quanto prima lei, Ministro, ci avesse portato un chiarimento parlamentare sulle dimissioni (ormai di una settimana fa) di un vertice dell'amministrazione Altrimenti le polemiche sul decreto segretato o no avvengono in un contesto di antiparlamentarismo che lascia francamente da solo quel richiamo, che la onora, ad evitare ogni miraggio di «radiose giornate». non sono arrivato in Aula con un testo già preparato in precedenza, perché volevo capire dalle sue parole quale poteva essere il ragionamento da sviluppare in questa sede e da condividere con i colleghi.

rallegrati, per quanto possibile in momenti così tristi e drammatici, per Pollicardo e Calcagno. Lei ha detto che il Copasir è stato aggiornato costantemente e lo sarà anche nelle prossime settimane.

ma che non è completa: i passaggi più importanti sono ancora da comprendere, da individuare e rappresentare all'interno di un organismo che è chiamato ad affrontare tematiche così delicate e che lo fa voglio dirlo a quest'Assemblea, perché è merito di tutti - in modo molto composto e serio. E lo fa perché ha costruito anche un certo tipo di rapporto

che rimangono ancora da chiarire vengano chiarite al più presto. Quest'oggi avremo l'audizione del ministro Pinotti e la settimana prossima verrà lei e verrà il direttore dell'Agenzia per i servizi esterni. In quell'occasione (non fra tre

deve essere sempre ritenuto importante, anche se qualcuno dirà che non è più urgente. Una cosa è l'urgenza e una cosa è l'importanza. Lei ha giustamente sottolineato le le modalità penose del rientro delle spoglie dei nostri due poveri connazionali. Forse questo è un altro dei punti su cui riflettere.

che sostanzialmente hanno indossato una divisa perché l'hanno trovata, e che hanno detto «da oggi comandiamo noi». E da qui deriva la loro inaffidabilità,

che ha già detto chiaramente che non vuole il Governo di unità nazionale. Del resto, sappiamo che quello di Tobruk, quello che noi riconosciamo e che la comunità internazionale riconosce, è un Governo

Questa realtà dovrebbe farvi comprendere come sia complicato, e forse anche inutile, cercare di addivenire

non siamo nel 1914, siamo nel 2016. Sono passati cento anni e la storia ci deve insegnare molto. Ci deve insegnare che certe situazioni vanno valutate attentamente e determinate scelte vanno assunte ben

concordo sull'utilizzo delle forze speciali in certe situazioni di emergenza all'estero, perché è l'unica soluzione per poter fare azioni propedeutiche alla messa in sicurezza di determinati luoghi. Non l'abbiamo ancora fatto,

mentre quella dell'impiego dei militari è necessariamente una scelta che deve essere fatta non comunicandola al Comitato ma condividendola a livello parlamentare. E su questo credo siamo tutti d'accordo. È necessario, quindi, capire che la situazione in Libia,

Parlavamo prima di storia con riferimento al 1914. Facciamo un salto un po' meno lungo nel passato e pensiamo - ad esempio - a quanto è accaduto, sottovalutando la presenza dei primi nuclei di al-Qaeda, una ventina di anni fa,

utilizzo un termine diverso - tollerata per un periodo troppo lungo, per un periodo drammaticamente lungo.

che i numeri che lei ha citato possono essere affrontati e sconfitti se effettivamente si interviene in tempi rapidi di comunità occidentali. Lo ripeto e lo ribadisco. Ma bisogna farlo, perché i 5.000 diventeranno, probabilmente, in tre mesi 10.000 e in sei mesi 20.000.

Noi non vogliamo a tutti i costi intervenire perché ci piace la guerra. Noi siamo preoccupati di ciò che potrebbe accadere nel nostro Paese e in tutto il mondo occidentale se non si interviene. È questo il vero problema. Se non si interviene, infatti, non è detto che, automaticamente, il nostro Paese sia tranquillo e si possano escludere eventuali atti terroristici nei nostri confronti. È tutto l'Occidente ad essere nel mirino. Quindi, non è con il non intervenire che ci si mette la coscienza a posto. Se non si interviene, però, si dà la possibilità all'ISIS di crescere in quelle zone. Si dà la possibilità all'ISIS di fare la tratta degli esseri umani. Si dà la possibilità all'ISIS di minacciare e ammazzare tanti cittadini inermi, che nulla hanno a che fare con la guerra, anche se è una guerra diversa (tanti, infatti,

una ulteriore destabilizzazione della Libia, che vorrebbe dire non avere più neanche il controllo di certe situazioni, oggi ancora sotto controllo, e di autorità vere; un ulteriore incremento dei flussi migratori verso il nostro Paese;

non conosciamo. Dovete fare qualcosa subito, condividendolo con il Parlamento. La rapidità della scelta è fondamentale per ottenere il miglior risultato possibile.

al debutto del suo dire, e cioè la necessità che il Parlamento, su questioni di politica estera, sostenga il Governo. di ciò convinto e lo ritengo, addirittura, quasi una sorta di premessa morale nella leale collaborazione tra le istituzioni di questo Paese.

Governo: cosa il Governo italiano vuole e quali precisi impegni internazionali ha assunto nei confronti degli alleati. Signor Ministro, lei mi dovrà concedere che non è apparso del tutto usuale il modo di rapportarsi a noi, al Paese Italia e al Governo italiano, utilizzato da alcuni alleati. Io non ricordo, non ho memoria

E non mi si venga a dire che ha trovato questo del tutto legittimo e incontrovertibilmente chiaro anche il Governo italiano. Perché si è dimesso il segretario generale della Farnesina? Che cosa sta accadendo nei rapporti tra noi e i nostri alleati?

Mi perdoni, signor Ministro, ma gli scenari che vengono disegnati non solo dagli alleati, ma anche da punti di riferimento per la nostra riflessione sulla nostra cultura di difesa, come il generale Vincenzo Camporini, ad oggi membro dell'Istituto affari internazionali e uomo di punta della storia recente della nostra difesa, dicono tutt'altro. Dipingono una Libia già tripartita, dove operano, in uno scenario internazionale complesso, gli alleati con precisi riferimenti a territori regionalizzati, (la Tripolitania, la Cirenaica e il Fezzan): i francesi vengono su dal Mali gli angloamericani in stretto rapporto con al-Sisi e l'Egitto. E noi che ruolo abbiamo? Qual è il nostro ruolo? Quali impegni abbiamo assunto? Mi si perdoni l'ironia, ma non vorrei che qualcuno, nella convinzione presuntuosa di masticare l'inglese più degli altri, si sia trattenuto con il presidente Obama qualche minuto di più senza interprete e abbia pronunciato qualche «*Yes, of course*» di troppo

Ed è desolante vedere lei abbandonato da questo Governo, solo in quest'Aula, perché anche il Ministro della difesa si è prontamente allontanato per non essere rampognato sull'essenziale. Ma come si fa a parlare in un'intervista di 5.000 uomini. 5.000 cosa? Se esistono piani dei nostri Stati Maggiori per i nostri impegni internazionali, non devono diventare oggetto di interviste. Vorrei che lei, signor Ministro, comprendesse che questo Parlamento vuole difendere il suo Ministro degli affari esteri, vuole schierarsi a fianco del Governo nelle questioni che riguardano la politica estera. Per questo ci vuole un puntuale monitoraggio, attraverso l'attività parlamentare, di ciò che il Governo reputa opportuno. Certo, lei fa bene a rivendicare il principio di una doverosa azione politica che allontani gli avventurismi di natura militare. Ma proprio perché dobbiamo svolgere un'azione politica, dobbiamo avere chiari quali sono i contorni. Che cosa vuole dire che 28 brigate si combattono in Libia? Qual è il nostro ruolo? Mi si perdoni, ma siccome il Governo precedente ha fatto attività di formazione dell'esercito libico, appoggiandosi a quelli che oggi stanno a Tobruk, come si fa ad immaginare che il nostro impiego sarà

il Governo non ha ancora chiarito nulla, non ha ancora detto che veramente sarà così. E proprio per questo, per un Parlamento che vuole aiutare il suo Governo è indispensabile comprendere - se possibile, non nel salotto di una *soubrette

Quali sono gli impegni assunti ieri nel vertice di Venezia con l'alleato francese, che invece in Libia si sente ancor più con le mani libere? Io credo che questi sommessi richiami possano essere utili al Governo per rafforzare la propria posizione, per mantenere un comportamento lineare nelle relazioni con il Parlamento, con l'obiettivo di essere utile al nostro Paese, di perseguire l'interesse nazionale e uno scopo di pace generale attraverso il quale noi intendiamo ricoprire fino in fondo il nostro ruolo di alleati affidabili. *(Applausi Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la crisi della Libia coinvolge l'Italia da vicino. Ci sono ragioni storiche, culturali, politiche ed economiche a dirlo e, quindi, a chiamare in causa il nostro Paese. Non ho citato - e lo sottolineo - ragioni di tipo militare, semplicemente perché qualsiasi intervento in tal senso andrebbe ponderato in ogni minimo dettaglio e, certamente, nel contesto della comunità internazionale. Signor Ministro, abbiamo apprezzato alcune sue recenti dichiarazioni sulla Libia, in particolare quando lei ha detto chiaramente che, prima di qualsiasi intervento mirato, e solo su richiesta di un Governo libico legittimo, serve che la Libia riesca a far vivere, non solo nei numeri, una coalizione unitaria in grado di stabilizzare il Paese. Il dramma dell'instabilità prodottasi in Libia dopo la caduta di Gheddafi ha in parte disintegrato la Libia. Dobbiamo certo riflettere sui molti errori compiuti - in verità non solo in Libia - dall'Occidente durante la fase delle cosiddette primavere arabe. Chi parla in questo momento ha assunto in passato posizioni estremamente critiche, anche con riguardo all'azione di un'Europa che, forse senza la necessaria dose di riflessione, ha assecondato azioni (politiche e non solo) poi poi rivelatesi avventate, in Libia e in altri scenari della tormentata area nordafricana e mediorientale. Ma recriminare sul passato non serve. Dobbiamo oggi riflettere - e il dialogo tra Governo e Parlamento, che deve essere costante e continuo, è essenziale - su cosa fare per stabilizzare la Libia nella cornice della legalità internazionale. Qualche commentatore ha evocato la necessità di una sorta di riedizione del Piano Marshall, con cui poter sostenere la rinascita economica e istituzionale della Libia, e non solo. Fare generalizzazioni è insidioso e certamente le condizioni storiche e politiche di oggi sono diverse da quelle dell'Europa uscita dalla guerra settant'anni fa. Tuttavia, ritengo che il principio sia giusto: impegnare le potenze occidentali in un progetto di sostegno e di nuovo sviluppo a favore di aree assolutamente strategiche sotto molti punti di vista per il mondo intero. per il mondo intero. Naturalmente non si tratterebbe di un impegno facile, né dagli esiti scontati. In Libia, oggi, è fortemente presente il terrorismo fondamentalista dello Stato islamico. La Libia è anche la terra promessa per le miriadi di trafficanti di esseri umani. Ci troviamo, in altre parole, di fronte a un Paese sull'orlo del baratro, in cui circolano più armi che persone, ma con il non secondario particolare che al suo interno vi sono forze politiche e militari che hanno interesse a che questo baratro sia irrimediabile e che la Libia rimanga in uno stato di caos. in un contesto tanto difficile, bisogna ponderare ogni passo e non cedere alla tentazione dell'avventurismo. In tal senso il Gruppo AL-A condivide quanto affermato in un'intervista di qualche giorno fa dal Presidente del Consiglio: un intervento di supporto militare in Libia dipenderà dalle richieste del Governo libico e da una risoluzione delle Nazioni Unite. Questa è un'esigenza imposta dall'appartenenza dell'Italia alla comunità internazionale e anche - mi permetto di dire dalla logica constatazione che, quando si interviene militarmente, bisogna pensare alle conseguenze non solo nel breve periodo. Molte esperienze del passato, anche recente, ci insegnano che questa è la linea da seguire. Detto questo, l'Italia non può rimanere inerte di fronte al disastro che si sta consumando a poche centinaia di chilometri dalle sue coste meridionali. La prospettiva che si apre di fronte a noi è certo complessa. La vicenda drammatica dei cittadini italiani rapiti in Libia - a tal proposito desidero esprimere in questa sede i sensi del nostro cordoglio alle famiglie delle due vittime, Fausto Piano e Salvatore Failla - è stata lo specchio del caos che avvolge un Paese ormai senza Stato dalla fine di Gheddafi, in balia di milizie, tribù, bande criminali e jihadisti, che si contendono il territorio e sfruttano gli ostaggi stranieri per finalità di riscatto o per ottenere una legittimazione politica. Proprio le autorità di Sabrata (città nella quale, la settimana scorsa, hanno avuto luogo violenti scontri armati tra islamisti e milizie), che hanno avuto in custodia gli italiani, rivendicano la propria autonomia da Tripoli e vogliono essere considerate un interlocutore forte per i futuri assetti della Libia. Impegnarsi per la stabilizzazione di questo Paese è un compito arduo che non può prescindere da un complesso lavoro di dialogo e trattativa con i diversi poteri politici che controllano parti del Paese e con i poteri tribali che, dopo la caduta del regime di Gheddafi, sono tornati prepotentemente sulla scena. Infine, colleghi, riteniamo che l'azione dell'Italia, grazie alla sua posizione geografica nel centro del Mediterraneo e al suo ruolo storico e culturale nella regione, debba anche svilupparsi con sempre più forza sul piano diplomatico per avere un maggiore e più convinto impegno sulla crisi libica da parte di attori, sovranazionali e nazionali, che sono parte dello scacchiere geopolitico della crisi, ma che finora, anzitutto a causa di forti instabilità interne e delicate dinamiche internazionali, hanno avuto un ruolo oggettivamente non deciso. Mi riferisco, in primo luogo, alla Lega araba e all'Unione africana, entrambe organizzazioni internazionali cui la Libia tuttora aderisce, ma anche a vari Paesi nordafricani e mediorientali. L'Europa, gli Stati Uniti e la Russia sono oggi in prima fila e ciò è normale. C'è davvero bisogno di una forte cooperazione anche su altri fronti

La crisi politica e militare della Libia è, infatti, anche di carattere sociale e sanitario e, in ultima istanza, potrebbe portare a sempre maggiori flussi migratori verso le nostre coste. l'altro ieri è intervenuto su questo aspetto dall'Algeria, dove si trovava in visita, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, secondo cui «Se sul piano politico non vi saranno dei progressi, la crisi umanitaria in Libia si aggraverà e così le minacce alla sicurezza, compresi gli attacchi dello Stato islamico». Signor Ministro, il Gruppo parlamentare AL-A valuta in modo positivo le dichiarazioni e i passi finora sostenuti dal Governo. L'Italia non può e non deve voltarsi dall'altra parte rispetto a quanto sta avvenendo in Libia. Dobbiamo, quindi, muoverci nel quadro della comunità internazionale ai livelli che saranno necessari. Signor Ministro, ha detto bene: fermezza, prudenza, responsabilità. È questa la

Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei anzitutto dare atto al Ministro degli affari esteri di alcune importanti puntualizzazioni che ci ha offerto questa mattina, divenute a mio avviso necessarie e, anzi, urgenti, visti i non lievi equivoci determinatisi nelle ultime settimane per quanto riguarda la situazione in Libia e anche le responsabilità, i compiti e gli intenti dell'Italia.

di informazione utili e si è riservato di darcene altri, essendoci ancora non poco da scavare in quella vicenda. Soprattutto,

un gravissimo problema per la comunità internazionale, come sappiamo. È un problema da affrontare su molti fronti - non solo su quello libico - e su molteplici versanti, e non solo su quello militare.

il crollo di ogni forma di legittimazione statuale in Libia. Parlo appunto della strategia dell'ISIS, della presenza e dell'insediamento dell'ISIS in Libia e anche di una sua possibilità di consolidamento e di ulteriore espansione.

la Libia. Siamo virtualmente partecipi di una vasta coalizione che si sta delineando nei confronti del fondamentalismo islamico, delle sue minacce e anche della sua presunta aggregazione statuale. Bisognerà concordare con gli alleati in che misura l'Italia debba farsi partecipe su tutti i fronti secondo le necessità del contrasto al fondamentalismo, al terrorismo e all'ISIS in Libia e altrove. Quando si è parlato - quotidianamente da qualche settimana - di una missione in Libia a guida italiana, ruolo che il Governo ha rivendicato e che è stato comprensibilmente stato comprensibilmente orgoglioso di essersi visto riconoscere dagli alleati, certamente non si parlava di una missione militare contro l'ISIS. Non se ne parlava un anno fa perché non c'era ancora questa presenza insidiosa

sarebbe grottesco pensare che ci possa essere una lotta all'ISIS su tanti fronti e in tante situazioni diverse a guida italiana.

legittimo capace di preservare l'integrità territoriale della Libia e di salvaguardare le sue potenzialità di sviluppo, fondate in larga misura sulle risorse energetiche. Comunque, per questa missione, che può prevedere alcuni impieghi limitati di reparti speciali, oltre che di servizi di sicurezza, come si è largamente detto e scritto, il Governo, comprensibilmente, ritiene indispensabile che si realizzino alcune condizioni

Dal momento che si torna talvolta a parlare piuttosto a vanvera dell'intervento NATO in Libia su mandato delle Nazioni Unite nel 2011, vorrei ricordare che allora ci fu legittimazione o, anzi, iniziativa internazionale delle Nazioni Unite; e ci fu l'approvazione del nostro Parlamento nelle sedute del 23 e 24 marzo 2011 con l'approvazione a larghissima maggioranza - compreso il Partito Democratico, allora all'opposizione - di quelle mozioni. L'unica cosa che nel 2011 non potevamo certo attendere è che ci fosse una richiesta del Governo libico, dato che il mandato delle Nazioni Unite era rivolto a colpire

abbiamo un grande punto interrogativo che è il se, quando e come si formerà un nuovo Governo nazionale unitario che richieda l'aiuto dell'Italia. Purtroppo molte nostre attese sono state deluse. Ieri sembra che il Presidente del Consiglio abbia detto che non c'è un tempo infinito per la costituzione di questo Governo, usando una frase secondo me del tutto comprensibile, anche se un po' criptica. In attesa che si compiano le condizioni necessarie noi facciamo comunque quello che possiamo, già ora in Libia, specialmente sul piano umanitario. Altra cosa è, appunto,

fare molta attenzione a minacce dirette per l'Italia e ipoteticamente per il suolo italiano. È sacrosanto il richiamo all'articolo 52 della Costituzione, ma noi dobbiamo anche tenere presente che c'è già una copertura internazionale (ed è prevedibile che ci sia ulteriormente) sulla base di quel famoso Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (che credo pochissimi abbiano avuto, anche tra quelli che scrivono sui giornali, l'avventura di leggere). non dimentichiamolo, segnando una differenza radicale rispetto all'operato della Società delle Nazioni, quando c'erano il fascismo e il nazismo in ascesa, prevede (è

violazioni e minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. Quindi, quello è il quadro in cui si inscrive la ben più generale questione del confronto con le minacce del fondamentalismo islamico e con la guerra e con la guerra scatenata dall'ISIS. Naturalmente tutto questo va fatto nell'ambito delle nostre possibilità e di una giusta ripartizione di compiti con i nostri alleati, all'interno - ripeto - della vastissima coalizione che si delinea. Certo,

italiani forse è venuta in mente improvvidamente all'ambasciatore degli Stati Uniti pensando a quello che è stato il nostro impegno in Afghanistan, perché in Afghanistan il nostro impegno ha sfiorato le 5.000 unità, le 5.000 unità, schierate sul campo in condizioni molto difficili. Vorrei dire soltanto, se mi è permesso, che ho vissuto, insieme con alcuni colleghi che erano già in Parlamento nelle precedenti legislature, legislature, i momenti più dolorosi della mia esperienza di Presidente della Repubblica recandomi a Ciampino ad accogliere le salme dei nostri caduti in Afghanistan, abbracciando i loro familiari e onorando il loro sacrificio nelle grandi

qualcosa di contrario ai nostri riferimenti storici, ideali e culturali il ricorso alle armi nei casi previsti dallo Statuto delle Nazioni Unite. Generare Unite. Generare l'illusione che non avremo mai, nel nostro futuro, necessità di interventi con le nostre Forze armate, in un mondo che ribolle di conflitti, di tensioni e di gravissime minacce, sarebbe veramente ingannare l'opinione pubblica, sollecitare un pacifismo di vecchissimo stampo, che non ha ragion d'essere nel mondo d'oggi e già nel mondo quale era uscito dalla Seconda guerra mondiale. Onorevole Ministro, mi auguro che questi chiarimenti servano a ben evitare ulteriori equivoci e a prepararci a quello che dobbiamo fare, nei nostri limiti, con grande senso di ponderazione e di responsabilità, in Libia, per la stabilizzazione della Libia, e in generale - in Libia e altrove - per contrastare l'offensiva del fondamentalismo islamico. *(Applausi

necessario affermare, con nettezza e con forza, da parte nostra, che quello che è accaduto nell'ultima settimana e in questi ultimi giorni non è accettabile e spero davvero non si verifichi

abbiamo compreso che qualcosa di grande si stava muovendo e che i tamburi di guerra, che lei stesso ha citato, avevano iniziato a rullare principalmente dai titoli della stampa internazionale, dalle interviste e dalle precisazioni dell'ambasciatore degli Stati Uniti e anche dalle dichiarazioni televisive del nostro Presidente del Consiglio e di vari Ministri, perché almeno fino ad oggi nessuno ha avvertito l'obbligo di portare tempestivamente qui, nell'unica sede propria, questa discussione. nemmeno dinanzi al fatto che agenti dei nostri servizi operano in territorio libico e che droni americani partono dalla base di Sigonella per bombardare le postazioni del Daesh in Cirenaica, come è stato ricordato; neppure nel caso della pagina drammatica costituita dalla tragedia degli ostaggi: quest'ultimo punto, almeno fino ad ora, il Governo aveva sentito il bisogno di dire qualcosa di più preciso, nella sede più appropriata. Insisto, questa è l'unica sede possibile nella quale avviare una discussione

senza poter votare e avere una voce in capitolo, definitiva e concreta, su un tema come questo, ci sembra, in una vicenda così complessa e delicata, un punto che, se fossimo al Governo, non sottovaluteremmo con tanta semplicità. Il presidente Renzi ha affermato qualche giorno fa, da un salotto televisivo, che se ci sarà un intervento militare, esso dovrà essere prima approvato dal Parlamento. Vorrei dire con chiarezza al Presidente del Consiglio e anche al Ministro che questa non è una gentile concessione,

al Parlamento bisogna rivolgersi non soltanto a cose fatte o ad accordi già presi, magari con le truppe sul punto di imbarcarsi, ma il Parlamento deve sapere

limitate, che grazie ad una modifica approvata in fretta e furia, in un clima molto particolare, come quello seguito alla tragedia di Parigi, consente oggi al Governo di avere facoltà di decidere in autonomia, senza il controllo parlamentare e soltanto con l'obbligo di informare il Copasir. A maggior ragione, quando scelte di questo genere si configurano come atti di guerra o che possono preparare il terreno

la scena politica e pur non essendosi fatto travolgere da isterie belliche, vorremmo anche dire con grande nettezza che noi non riteniamo sufficienti le rassicurazioni del Presidente del Consiglio.

ma anche perché le stesse dichiarazioni rese dal presidente Renzi anche ieri a margine o durante l'incontro con il presidente Hollande ci sembrano probabilmente leggermente, ma comunque diverse da quelle rese nei giorni precedenti. Per esempio, la richiamata condizione imprescindibile di un Governo unitario libico ieri è diventata una condizione auspicabile. Come voi capite bene - e mi rivolgo ai membri del Governo su una vicenda delicata come questa le parole non sono semplicemente importanti, ma evidentemente sono decisive. Pertanto, anche quando si cambia un aggettivo o un verbo,

che in queste ore sia in corso un'intensa attività diplomatica, probabilmente una vera e propria trattativa, con l'obiettivo di dar corpo ad una spedizione internazionale, la cui guida, il cui peso e la cui responsabilità ricadrebbero soprattutto sul nostro Paese. Vorrei quindi dire in maniera inequivocabile, in modo che perlomeno resti agli atti di questa discussione parlamentare, che a nostro avviso sarebbe un errore gravissimo, esiziale. una missione in Libia finirebbe per avere gli stessi effetti disastrosi di quell'indifendibile 2011, di cui sono ovviamente responsabili anche quelle stesse forze politiche di destra

generale che condusse a quel drammatico errore, a quello sciagurato intervento militare che purtroppo ha soltanto avvantaggiato il crescere in tutti questi mesi e anni del fondamentalismo islamico e non ha minimamente risolto risolto il caos di quell'area, aggravando una condizione politica già difficilissima e determinando la situazione disastrosa alla quale ci siamo dovuti riferire nei mesi e negli anni successivi. Noi pensiamo che a pagare i prezzi sarebbero, ancora una volta, i più deboli, quella popolazione libica già massacrata da anni di guerra per bande. Pensiamo, invece, come abbiamo detto tante volte in queste settimane, che l'impegno dell'Italia e dell'Unione europea debba essere profondamente indirizzato a raggiungere l'accordo per la costituzione di un Governo unitario capace di avviare un processo di pacificazione. Naturalmente i costi di una simile spedizione

che l'intervento militare è certamente escluso, almeno in assenza di una richiesta di un Governo unitario libico, però legittimato dal consenso elettorale e non un semplice fantoccio; deve affermare con altrettanta chiarezza che un qualunque intervento, anche il più limitato, non è neppure immaginabile fuori dal quadro di una legittimazione internazionale delle Nazioni Unite e privo delle caratteristiche di una vera missione internazionale e non di un impegno essenzialmente essenzialmente italiano. Senza queste condizioni preliminari, signor Presidente, crediamo che un eventuale impegno italiano non possa nemmeno essere preso in considerazione. Vorremmo anche aggiungere che, pure in presenza di queste eventuali condizioni (oggi peraltro molto lontane), crediamo in ogni caso che sarebbe molto rischiosa e molto pericolosa un'impresa i cui esiti potrebbero essere molto seri e molto

In questo caso non si tratta semplicemente di rivendicare una scelta pacifista, che pure - vorrei ricordarlo - è patrimonio non del mio Gruppo parlamentare, ma della nostra Costituzione e della nostra Repubblica*. (Applausi dal Gruppo con realismo e con efficacia (tutto il contrario dell'ideologia) in uno scenario complesso, consapevoli della possibilità concreta di rafforzare il Daesh molto più che di indebolirlo, come peraltro sostiene la stragrande maggioranza

ebbene, credo che ripetere quell'errore oggi, tanti anni dopo, sarebbe davvero una scelta drammatica, che non avrebbe alcuna giustificazione.

le parole del ministro Gentiloni Silveri, a mio avviso, sono state convincenti; i rilievi nei confronti del Governo incerti, confusi, contraddittori. Non ho ben capito - confesso ai colleghi dell'opposizione - alcuni rilievi che sono stati mossi, che francamente mi sembrano lunari: la tempestività nelle comunicazioni del Governo dopo la tragedia dei nostri due cittadini, cittadini, Failla e Piano, che ancora, in questo momento, aspettiamo di riavere, seppure privi di vita, sul territorio nazionale. cosa avrebbe dovuto fare il Governo? Mentre altri due connazionali dovevano essere recuperati e salvati, da operazioni anche coperte (mi auguro che siano così), doveva forse venire in questa sede e dilungarsi sui particolari, compromettendo o rischiando di compromettere la vita dei due italiani ancora vivi in Libia? Mi sembra che sia una cosa che contrasta il buonsenso, senza bisogno che io sprechi altre parole. Che cosa doveva fare il Governo in riferimento ad altre vicende? Qualcuno esprime dei rilievi sul fatto che ci possano forse essere persone riconducibili ai servizi d'informazione e ai servizi segreti italiani in territorio libico. C'è una copertura, diciamo così, in termini di dispositivo che consente al Governo di fare questo. Ma vogliamo prenderci in giro? Con quello che sta capitando in Libia, noi saremmo più tranquilli se l'Italia non avesse alcuni "sensori" che operano in quel Paese per capire cosa sta accadendo e prevenire quello che può capitare? Ma scusate, siamo sulla luna se pensiamo questo. Non abbiamo capito nulla di ciò che sta capitando nel mondo dove, come giustamente ha detto il ministro Gentiloni Silveri richiamando le parole di Obama, peggio degli Stati canaglia ci sono solo gli Stati dissolti. allora in questa situazione. E poi, scusate, poiché io da oppositore, in tutti i passaggi della mia vita parlamentare, ho sostenuto la politica estera di Governi diversi, anche quando quei Governi avevano il mio voto contrario, vi prego di non usare l'ipocrisia che ho sentito oggi da parte di chi, dopo essersi scatenato nelle più violente e inconsulte critiche nei confronti del Governo dice

Noi oggi siamo tutti impegnati, in Parlamento come al Governo, per rivendicare un ruolo di guida per l'Italia in quello che può essere il futuro della Libia. Questo cosa significa? Questo coincide con il fatto che vogliamo inviare in Libia migliaia di uomini? Ma in base a che cosa? Il ruolo di guida si esplicita anche nell'indicare agli alleati le questioni che noi vediamo meglio di loro. La questione che vediamo meglio di loro è una ed è semplice: se noi vogliamo

schierare migliaia di militari in campo. Mandiamo allo sbaraglio migliaia di persone e realizziamo immediatamente una contrapposizione tra tutti i libici e la comunità occidentale;

voglio parlare di ciò che lei ha appena detto: non in nome di un astratto principio di pacifismo perché con le bandiere della pace non si batte il terrorismo. Quando siamo andati in

E infatti, a qualche anno di distanza, abbiamo pacificato i Balcani e oggi i Paesi che ne fanno parte bussano alla porta dell'Unione europea e sono parte del nostro sviluppo futuro. Santangelo)*. Quando in Italia si è fatta la resistenza contro i nazisti, non si è fatta con la bandiera della pace. Leggete la storia se non lo sapete!

Il punto che vorrei evidenziare, e lo ha detto molto bene il presidente Napolitano,

da posizioni politiche antitetiche abbiano avuto la stessa posizione sulla Libia. Evidentemente questa posizione, come ha giustamente detto il presidente Napolitano, è una posizione di ragionevolezza e di responsabilità, che noi siamo convinti per il momento richieda un interlocutore obbligato, che è il Governo costituitosi sotto l'egida dell'ONU. Poi, certo, quel Governo andrà aiutato. Se dovrà entrare a Tripoli, perché non potrà governare dall'estero, noi dovremo impiegare tutte le energie nel modo e nella forma che il Governo riterrà opportuno e che verrà a proporre in Parlamento. Ma questa è la metodologia, e non è forma: questa è sostanza di politica estera. Vorrei poi illustrare altri tre punti. La prima riguarda la tripartizione della Libia. Libia. Io non credo affatto che la tripartizione della Libia sia già stata sancita, come qualcuno, facendo l'informato, è venuto a spiegarci. La tripartizione della Libia non c'è ancora. qualcosa ci induce ad avere una preoccupazione che aumenta. Voglio essere esplicito. Noi tutti che la comunità dei Paesi mediterranei (a partire dall'Egitto e a seguire l'Italia, la Francia e tutti gli altri) sostiene la mediazione dell'ONU e di Kobler. Sappiamo anche che l'Egitto ha un rapporto particolare con il generale Haftar.

allora qualcosa che non torna. Se l'Egitto fosse così impegnato a garantire l'unità libica, il generale Haftar non sarebbe probabilmente in condizioni di muoversi con questa spregiudicatezza. che pensi che la tripartizione possa essere una soluzione, è un'evenienza, ministro Gentiloni Silveri, che lei senz'altro avrà valutato, ma che è da vedere con grandissima preoccupazione. A tal riguardo, io ho una grandissima preoccupazione, perché, così come sarebbe dissennata oggi un'azione militare di massa

dello Stato un ambasciatore di primissima qualità, che ha servito il Paese con serietà, che si è rapportato al Parlamento con grande rispetto istituzionale dei ruoli reciproci. È dunque giusto che dal Parlamento

Io l'ho sollecitata pubblicamente. Naturalmente, poiché sono un uomo delle istituzioni, penso che la scelta non spetti al Presidente della Commissione affari esteri ma al Governo. Pertanto, ciascuno faccia il suo lavoro. Voi fate il vostro, e noi vi controlleremo.

contraddittorie. Chiaramente, in molte circostanze coincidono con il tentativo di prendere tempo; non è qualcosa su cui possiamo transigere, perché dietro Regeni c'è il decoro e la dignità di una Nazione e la difesa della vita umana e dei nostri concittadini. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli cittadini che ci ascoltate (fortunatamente ci ascoltate, perché quanto detto in alcuni interventi è assolutamente inaccettabile), parlare di bombe di pace è una bestemmia

di esprimersi su strategie che riguardano la vita di tutti noi italiani. Ciò che è stato raccontato da lei, signor Ministro, è elementare e non basta assolutamente.

dell'Italia in politica estera e di difesa non viene più fatta in Parlamento, non viene più fatta nemmeno da questo Governo di burattini: viene fatta dagli Stati Uniti d'America, oggi più di ieri, e questa cosa è assolutamente inaccettabile. La vera realtà non è quella che è stata descritta dal ministro Gentiloni. ci sono degli interessi economici che vanno al di sopra di tutti gli altri interessi. Andiamo a vedere che cosa ha già deciso questo Governo con dei cavilli legislativi. Il Primo Ministro ha già dato facoltà agli Stati Uniti di dispiegare dei veicoli armati che partono dalla Sicilia:

l'articolo 78 della Costituzione, dove si dice che qualsiasi azione di guerra deve essere stabilita, ragionata e votata in Parlamento, e non da Renzi né dal suo Governo. Le ricordo l'articolo 11 della Costituzione in tutte le sue parti, anche la seconda. Quando si dice che l'Italia sarà a capo di una fantomatica azione in Libia, ma da chi è stato deciso?

ma quest'ultimo non può essere mortificato soltanto come un ente ratificatore di quello che sta facendo un Governo che nemmeno gli italiani hanno più voluto. Questo Governo infatti è sostenuto da maggioranze che non sono state mandate qui dagli italiani; sono maggioranze che probabilmente Giorgio Napolitano ha voluto,

Signor Presidente, vorrei partire dalla conclusione del ministro Gentiloni, il quale ha terminato il suo intervento parlando di fermezza, di prudenza e di responsabilità. Sono concetti che condividiamo, ma che, a nostro avviso, devono essere declinati nel quadro della normativa internazionale che regola i rapporti fra gli Stati e le possibilità di intervento degli Stati in zone come quella libica. Giustamente, negli interventi che mi hanno preceduto, qualcuno ha ricordato l'articolo 11 della Costituzione. Lei, signor Ministro, ha ricordato l'articolo 52, secondo il quale è sacro dovere dei cittadini italiani difendere la patria. Ma noi ci troviamo in un contesto internazionale nel quale insistono la risoluzione n. 2259 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che in un passaggio

contro l'ISIL (cioè il Daesh, così come viene evocato) e contro altri gruppi terroristici presenti in Libia, in particolare Ansar al-Sharia (che giustamente, dice la risoluzione n. 2259, è collegato con al-Qaeda). Qualcuno stamattina ha ricordato anche il *Chapter VII* della Carta delle Nazioni Unite, che all'articolo 42 prevede, laddove le misure di blocco economico e militare di un'area non fossero sufficienti per risolvere il problema,

possono e debbono allora essere declinati anche nel quadro della normativa internazionale, che a mio avviso consente, anche al nostro Paese ed anche sotto la guida del nostro Paese, ai Paesi alleati di intervenire, laddove lo dovessero ritenere opportuno, nell'interesse del nostro Paese e nell'interesse della comunità occidentale. Ministro, devo dire che stamattina la parte più deludente del suo intervento è stata quella che io vorrei definire «il buco di Sabrata». Non ho capito cosa sia accaduto effettivamente ed ho l'impressione che su questo punto non siano state date risposte sufficienti. In primo perché i quattro tecnici italiani sono andati in automobile, su indicazione ed autorizzazione dell'azienda Bonatti? Avrebbero dovuto prendere una nave, sbarcare a Mellita ed avvicinarsi molto più agevolmente al posto di lavoro e non invece attraversare il confine libico là dove sono stati intercettati.

che ci dovrebbe essere in questi casi, necessaria e obbligatoria laddove ci siano degli ostaggi? Perché Sabrata o la polizia di Sabrata ha autorizzato l'intercettazione del convoglio? Perché la municipalità di Sabrata ha sequestrato le salme dei due poveri italiani ed ha sequestrato anche i due italiani

criminali del Daesh, cioè quaranta tunisini (nessun libico) e purtroppo anche due poveri ostaggi serbi. Quindi Sabrata non è un'area dove le cose si svolgono in una maniera riconoscibile ed intelligibile. Che ruolo ha avuto il Governo di Tripoli? Abbiamo assistito ad una strana ed inquietante conferenza stampa, dove c'era un silenzioso sindaco di Sabrata (presunto tale, ma immagino che lo sia), lo sia), il quale ci teneva tantissimo ad essere presente, dopo che la sua polizia ha ucciso due cittadini italiani, accompagnato da un Ministro degli affari esteri presunto del Governo di Tripoli, che rivendicava l'azione che guarda caso aveva portato al danno

di Salvatore Failla e Fausto Piano. Mi auguro che ciò sia vero e anche che non sia stato fatto scempio dei loro corpi durante le autopsie che il Governo di Tripoli ha ritenuto di fare, non so con quali autorizzazioni.

però l'impressione che la riservatezza dovuta (che, per senso di responsabilità, noi rispettiamo) non possa prescindere dalla ricerca della verità.

La sintesi avvenuta tra le tribù sunnite di Tikrit e il Daesh sta a dimostrare che là il Daesh è una forza anche politica, statuale e di organizzazione, che raccoglie le tasse ed applica la *shari'a*, ma che sicuramente rappresenta uno Stato. il Daesh è un'altra cosa. In quel Paese si tratta soprattutto di criminali (perché così vanno definiti) che vengono dall'esterno e non hanno trovato connivenze particolari con le tribù e le popolazioni siriane.

perché sembrava che fossero 200, 300, 400 coloro che dovevano attraverso la frontiera ed attaccare la città tunisina, mentre sono passati solamente in 60, la metà dei quali, grazie al cielo, sono morti, facendo vittime nella polizia municipale e vittime civili. Ciò vuol dire che

C'è quindi uno spazio per un intervento chirurgico mirato che vada ad attenuare e ammorbidire le difese di questi criminali. Di tutto questo non si parla. Sembra che stiamo parlando, per la prima volta, di operazioni militari che mi auguro esistano (infatti, quando sento dire che sono presenti agenti e servizi inglesi, francesi e americani, non si dice che sono presenti anche gli italiani). Quanto successo a Sabrata mi preoccupa perché non è una città di milioni di abitanti. È una città con poche migliaia di abitanti.

XVII)*. C'è qualcosa che non ha funzionato complessivamente in questa storia e su questo, caro Ministro, non abbiamo avuto alcun tipo di risposta. nel recente passato, soprattutto il Gruppo Movimento 5 Stelle, ha detto una cosa che ho condiviso: le guerre si vincono con azioni mirate, tipo quelle che ho cercato di immaginare, ma anche tagliando il cordone economico. al Daesh in Iraq e Siria fosse impedito il trasporto illegale di petrolio in Turchia e in altri Paesi confinanti, tutto sarebbe più semplice. In questa circostanza, abbiamo un caso simile:

non dico dei Governi perché è difficile riconoscerne uno che abbia legittimità internazionale. Si tratta di 67 miliardi che sono lì, ma gli stessi libici - una volta il rappresentante del Governo di Tobruk e una volta il rappresentante del Governo di Tripoli - partecipano ad assemblee di aziende italiane. Tra le aziende italiane c'è Finmeccanica. Noi abbiamo una tale contiguità e quantità di rapporti, anche di carattere economico e rilevanti, che consentono ad un rappresentante libico, in questo caso del Governo di Tripoli, di partecipare alle assemblee e di determinare con il proprio voto con il proprio voto il collegio sindacale. Ciò vuol dire che noi abbiamo una primazia nel rapporto con la Libia e tutti i meccanismi, statuali o no che siano di questo Paese, dovrebbero metterci in una condizione di assoluto privilegio di rapporto.

e ci riserveremo nell'ambito del Copasir di capire meglio quello che succede. Però, l'omissione di verità che questa mattina è stata fatta in questa avendo anche derubricato la comunicazione del Governo ad un'informativa e non avendo nemmeno dato la possibilità al Parlamento di votare su una mozione (cosa che, a mio avviso, sarebbe stata meglio per dare un'indicazione parlamentare), penso abbia oscurato e annebbiato ancora di più quello che è successo in questi tragici giorni.

Fausto Piano e Salvatore Failla e la nostra vicinanza alla loro famiglia. Bene ha fatto il ministro Gentiloni a confermare che il Governo italiano farà di tutto per accertare la verità sul sequestro dei dei quattro connazionali, la morte di Piano e Failla, così come sta facendo per accertare cos'è accaduto per l'orrenda uccisione di Giulio Regeni.

Ringrazio il ministro Gentiloni per la sua informativa e ne condivido l'analisi. Concordo con gli indirizzi di fondo del Governo italiano sulla questione libica: favorire la stabilizzazione politica e sociale della Libia; contenere l'emergenza terroristica; operare nella legalità internazionale e con il consenso delle autorità libiche. Sono noti i fatti - e non li ripeterò - gli errori, i ritardi e le omissioni che hanno determinato questa crisi. Dopo anni di deterioramento delle condizioni della Libia, ormai vastissime parti di quel Paese sono ridotte a laboratorio e base logistica per il terrorismo internazionale e per l'emigrazione clandestina. La Libia

con una realtà locale complessa e indecifrabile, uno scenario regionale denso di incognite, dove i tanti protagonisti fanno ciascuno il proprio gioco, alcuni pulito e altri sporco. Oggi, per la comunità internazionale, girare la testa dall'altra parte e non comprendere l'urgenza dei pericoli significherebbe trascurare il continuo aggravamento dell'instabilità di un Paese, che il terrorismo dell'ISIS vuole trasformare in una piattaforma, da cui far partire gli attacchi verso l'Italia e verso l'Europa. A cinque anni dalle rivolte di piazza, culminate con l'uccisione di Gheddafi, nonostante l'impegno delle Nazioni Unite e dei suoi inviati Bernardino Leon e Martin Kobler, non è stato sinora possibile insediare in Libia un Governo di accordo nazionale,

reparti armati dell'ISIS violano continuamente le frontiere con la Tunisia e hanno il controllo di 200 chilometri di costa e della città di Sirte, la mancanza del consenso di un Governo autorevole rende non praticabili le azioni necessarie alla stabilizzazione. In assenza della decisione di un Parlamento libico, che non c'è, qualsiasi intervento di questa o quella potenza occidentale verrebbe interpretato come una lesione della sovranità nazionale, irrigidirebbe le posizioni e alimenterebbe sentimenti antieuropei e antioccidentali. Conosciamo la molteplicità dei poteri locali, che si muovono autonomamente all'interno del territorio nazionale libico e sappiamo di dover valutare i rischi di una crescente presenza dell'ISIS e del suo controllo di parti sempre più ampie del territorio. Ieri è arrivato persino un nuovo attacco alle forze di sicurezza e dell'esercito tunisino - dell'esercito, addirittura! - in territorio tunisino, con scontri a fuoco e 55 morti. Consideriamo anche i forti interessi energetici italiani in Libia. l'energia non è soltanto un affare, ma è un bisogno, una necessità per l'Italia. Teniamo conto del ruolo che potrebbe essere attribuito all'Italia nell'opera di stabilizzazione. Per queste ragioni, condivido la posizione del presidente Renzi, quando dice che non è all'ordine del giorno la missione militare italiana in Libia, perché la prima cosa da fare è che ci sia un Governo solido, che abbia la possibilità di sollecitare un intervento della comunità internazionale e non faccia ripetere gli errori del passato. Il Governo italiano conferma, con queste parole, la gravità del pericolo e il nostro forte interesse per la stabilizzazione della Libia, ma tiene in debito conto i principi della legalità internazionale e le difficili condizioni di quel Paese. Per l'Italia, il rifiuto della guerra non è solo un precetto costituzionale. L'Italia - come ha detto prima il senatore De Cristofaro - è una Repubblica ancora giovane, che ha pagato prezzi molto alti alla violenza e alle guerre. Siamo però anche un popolo maturo, che sa distinguere tra l'aspirazione alla pace e la necessità di aiutare la costruzione di nuovi equilibri nell'Africa del Nord e nel Mediterraneo, e sa anche come deve difendere il proprio territorio nazionale e la vita degli italiani. Siamo un popolo che vuole capire il senso degli avvenimenti e cercare di prevederne le conseguenze. Gli italiani conoscono bene l'ipocrisia di una pace solamente declamata, retorica e predicatoria: la pace di chi non vuole vedere, né sa ascoltare. La storia ci ha insegnato che una pace che non viene difesa, cercata, conquistata, non produce pace, ma favorisce la guerra. Nella ricerca di una vera pace in un mondo devastato da decine di guerre locali, oggi l'Italia gode dell'autorevolezza internazionale conquistata con i risultati dell'azione delle sue Forze armate. Sono più di 5.000 i nostri soldati, aviatori, marinai impegnati a favorire la pace nel mondo. Ricordo questo dato per ringraziare le nostre Forze armate non solo per il loro impegno, ma ancora di più per la qualità e l'intelligenza del loro lavoro. Dobbiamo dare atto che è cresciuta in Italia una classe dirigente militare di assoluta lealtà democratica e di ottima qualificazione professionale. Le nostre Forze armate sono uno dei poli di eccellenza dell'apparato del nostro Stato la vastità dell'impegno internazionale delle Forze armate, dell'Italia conferma l'ampiezza e l'intensità delle situazioni di crisi che nel loro insieme stanno destabilizzando e insanguinando l'intera sponda Sud e Sud-Est del Mediterraneo.

I senatori del Partito Democratico apprezzano questo indirizzo e ringraziano il Governo per averlo reso pubblico. Concludo il mio intervento con poche considerazioni sulla fase che l'Italia, l'Europa, il Mediterraneo e l'intera comunità internazionale stanno attraversando. Mentre perdurano gli effetti di una crisi finanziaria che, a partire dal 2008, ha fermato gran parte dell'economia del pianeta, mentre i flussi migratori stanno assumendo dimensioni sempre meno controllabili, mentre la globalizzazione e le nuove tecnologie incidono in profondità nella stessa struttura delle Nazioni, mentre accade tutto questo, sempre più spesso nel mondo sentiamo analisti, commentatori, editorialisti e uomini politici pronunciare la parola «guerra». Guerra è una parola che gli italiani aborrano, che considerano estranea alle loro convinzioni e alla loro cultura, ma stiamo attenti. Il rifiuto della guerra non può e non deve impedirci di vedere quel che accade intorno a noi; non può oscurare l'abominio e la pericolosità del nuovo terrorismo internazionale, farci dimenticare la sua violenza estrema, la sua pratica di *kamikaze*, le sue esecuzioni rituali, la riduzione in schiavitù di donne, bambini e uomini, le minacce di distruzione assoluta della civiltà occidentale. Gran parte di quella che è stata autorevolmente definita una nuova guerra mondiale a pezzi ha origine proprio dalla violenza del nuovo terrorismo, dall'ampiezza del suo bacino di arruolamento, dalle sue disponibilità finanziarie, da forme organiche di complicità con le più spietate organizzazioni criminali. In questa difficile congiuntura, davanti a scenari internazionali così complessi, fa bene il Governo italiano a muoversi non solo con chiarezza di obiettivi, ma anche con molta attenzione e con grande cautela. Dobbiamo condividere fino in fondo una politica che che abbia chiara coscienza della gravità del pericolo, ma rifiuti l'avventura e ponga come propri obiettivi prioritari a qualunque decisione l'insediamento di un Governo libico unitario e rappresentativo, una chiara posizione delle Nazioni Unite, la presenza di una coalizione internazionale esplicita e solidale. Se per il nostro Paese queste sono le precondizioni di una seria politica a sostegno e di aiuto alla Libia, c'è qualcosa di più che noi senatori dobbiamo fare, che rientra nelle nostre responsabilità e costituisce un nostro primario dovere civile e politico. Ne ha parlato prima

entrando nel merito di decisioni che riguardano la nostra sicurezza nazionale e che attengono alla nostra politica estera e di difesa, è nostro dovere tener conto esclusivamente dell'interesse dell'Italia, del sacrificio delle nostre Forze armate e di sicurezza, degli obblighi che abbiamo contratto nei confronti dei nostri alleati internazionali. Nel tempo di maggior allarme per l'Italia dalla fine della Seconda guerra mondiale, sarebbe molto grave se ci facessimo prendere la mano dai nostri interessi particolari di partito o di schieramento, se prima che all'Italia pensassimo al nostro tornaconto elettorale o alle nostre tattiche parlamentari o usassimo dei non-argomenti, come ho sentito pronunciare dai senatori Lucidi e Santangelo. L'uso della politica estera e di difesa a fini interni significherebbe non solo tradire gli italiani, ma anche indebolire l'Italia sul piano internazionale e sottrarre alle nostre Forze armate e di sicurezza quel sostegno pieno e leale che è a loro dovuto dal Parlamento, senza distinzione tra destra e sinistra, tra antichi partiti e nuovi movimenti. Teniamo a mente che nelle grandi democrazie maggioranza e opposizione si contrappongono in tutto, ma mai quando è in gioco la sicurezza nazionale. Ricordiamocelo, perché è proprio su questo punto, sul valore unitario da dare alla difesa della Patria, che un Parlamento dimostra la propria maturità democratica.